colleghi, desidero rivolgere un commosso pensiero al ricordo del senatore Romualdo Coviello. Persona di fine cultura e rara sensibilità sensibilità politica, docente universitario stimato e apprezzato da colleghi e studenti, Romualdo Coviello è stato un instancabile protagonista della vita politica italiana e della Basilicata, oltre che un intelligente interprete delle istanze e delle potenzialità di quei territori. Una passione politica genuina fu la sua, coltivata con generosità e responsabilità sin dai primi incarichi che hanno visto intrecciare la sua carriera con la nascita del Consiglio regionale della Basilicata, di cui fu anche Presidente, oltre che assessore regionale all'agricoltura. Eletto per la prima volta al Senato nel 1987, tra le fila della Democrazia Cristiana, Romualdo Coviello è stato autorevole componente di questa Assemblea per ben cinque legislature e Presidente della Commissione bilancio durante la XIII legislatura. Ricordo gli anni che abbiamo condiviso tra i banchi di quest'Aula. Pur appartenendo a schieramenti contrapposti, Romualdo Coviello si è sempre dimostrato un avversario leale e dialogante, di cui non si potevano non ammirare l'onestà intellettuale, la ferma coerenza di pensiero, lo spirito concreto e pragmatico, l'inclinazione innovatrice, specie sul piano delle politiche pubbliche. un autentico uomo delle istituzioni e della democrazia, fermamente convinto che il confronto costruttivo e non lo scontro conflittuale fosse la strada maestra per tutelare diritti e aspettative dei cittadini. Un impegno, il suo, dedicato soprattutto al riscatto dei territori più fragili e deboli del nostro Paese e della Lucania in particolare, la sua amata terra che è sempre rimasta al centro della sua attività politica e per il cui sviluppo Romualdo Coviello non ha mai smesso di battersi, anche una volta conclusa la sua esperienza parlamentare. Nel rinnovare pertanto un sincero sentimento di vicinanza e cordoglio ai familiari, ai colleghi e agli amici del senatore Coviello, chiedo all'Aula di onorarne il ricordo osservando un minuto di silenzio.

Signor Presidente, lei ha usato le parole giuste per ricordare il senatore Coviello.

e lo hanno apprezzato. Romualdo Coviello aveva la capacità dello sguardo lungimirante

era un politico di razza, oltre che un economista competente e un meridionalista militante; un uomo grintoso, mai arrendevole, capace di convincere con una tenacia che non aveva eguali, mai doma. Era un uomo forte dei valori propri del cattolicesimo democratico dossettiano ed esponente di primo piano della Democrazia Cristiana lucana. un uomo che studiava, argomentava e conosceva il territorio come pochi altri. Con lui ho condiviso la gioia di una grande campagna elettorale,

di convincere gli elettori. Allora c'erano grandi temi nel dibattito lucano (il petrolio e il parco dell'Appennino) e una grande discussione, anche critica, tra i cittadini. Romualdo mi diceva di non temere, che bisognava avere capacità di ascolto di ascolto e convinzione dei cittadini attraverso gli argomenti giusti; quanto al petrolio, non tutto il petrolio, ma quello che poteva estrarsi dalla Basilicata in un quadro di sostenibilità e in un rapporto dignitoso con le compagnie petrolifere, mediato dallo Stato con un'intesa con le Regioni. E così avvenne. Quanto al parco, non il parco a tutti i costi, ma quello che difende i cittadini e lo sviluppo. Romualdo ci ha insegnato Il nostro ricordo è quindi intriso di affetto, stima e profonda gratitudine che io ho l'onore di esprimere a nome di tutto

Grazie a uomini come te possiamo dire che è falsa la solfa per cui tutta la politica e tutti i politici sono da gettar via. Ci sono stati donne e uomini che hanno fatto la politica con la p maiuscola e si ergono oggi come esempi per le nuove generazioni. Grazie Romualdo.

straordinario innovatore delle politiche agricole della Basilicata e, più in generale - come è stato appena ricordato dal collega Pittella un grande innovatore del Sud. È stato un protagonista indiscusso della nostra storia recente, proprio perché ha saputo mettere al servizio delle istituzioni il sapere e le conoscenze che gli arrivavano dal mondo accademico. Ha rappresentato nel migliore dei modi la comunità lucana e l'ha fatto anche a livello nazionale per molti anni, da senatore, non dimenticando le esigenze, le difficoltà, ma anche i punti di forza di una comunità così ricca come quella lucana. Sapere, studio, conoscenze, ma anche visione di lungo periodo e dialogo istituzionale sempre proficuo con tutti: sono le qualità che l'hanno reso un grande uomo politico, sempre attento alle preoccupazioni dei cittadini. Abbiamo avuto tutti modo di apprezzarne tutte le qualità umane, senza però tralasciare il suo contributo scientifico, professionale e civile, volto alla comune battaglia contro le diseguaglianze economiche e sociali, che ancora oggi purtroppo lacerano il nostro Paese. A nome del Gruppo Italia Viva-PSI ci uniamo al dolore della famiglia e della sua comunità. Lo ricordiamo come un uomo appassionato, da sempre in prima linea per correggere le storture del sistema e le disparità di una società che lui voleva più giusta e più equa. *(Applausi)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, anch'io intervengo a nome

e all'intera comunità lucana, alla quale Coviello ha dedicato la sua intera esistenza, prima in veste di ricercatore e studioso; poi di amministratore; infine, per molti anni, di senatore della Repubblica. Coviello - intellettuale, docente universitario, politico appassionato, meridionalista convinto - ha saputo coniugare, nei suoi ottantuno anni di vita, le sue diverse competenze e attività, convogliandole sempre verso il medesimo obiettivo: lo sviluppo della sua Regione, la Basilicata, e la modernizzazione e l'innovazione dell'agricoltura in una dimensione integrata con quella dell'intero Meridione. Ci piace ricordare il suo impegno in prima linea nei mesi difficili del *post* terremoto del 23 novembre del 1980, che colpì la Campania e la sua Basilicata. In quel momento Coviello, dopo essere stato ricercatore presso le università di Bari e della Basilicata, aveva scelto la politica attiva nella Regione Basilicata, rivestendo i ruoli di assessore all'agricoltura e alla programmazione economica e di Presidente dell'Assemblea regionale. Era un cattolico democratico d'ispirazione dossettiana, dunque estremamente sensibile e attento alla condizione delle aree socialmente e geograficamente più deboli e penalizzate del Paese; oggi diremmo sensibile alle diseguaglianze economiche, sociali e territoriali e alla necessità, ormai imprescindibile, di ridurle e, in prospettiva, sanarle. Nel 1987 fu eletto al Senato, dove sarebbe rimasto per quasi vent'anni come senatore della Democrazia Cristiana, poi del Partito Popolare, infine della Margherita; Presidente della Commissione bilancio tra il 1996 e il 2001. Al Senato il suo impegno rimase orientato nella stessa direzione: era convinto che la modernizzazione del Sud non dipendesse solo dall'industrializzazione, ma che il futuro della sua terra passasse anche e soprattutto per la modernizzazione del settore primario, dell'agricoltura. Crediamo che sia giusto concludere questo ricordo citando l'asse portante della sua riflessione di studioso e della sua attività di uomo politico: l'idea di uno sviluppo autopropulsivo centrato sulla programmazione non solo della Basilicata, ma dell'intero Mezzogiorno, senza assistenzialismo, ma anche senza localismi di sorta; in una dimensione integrata aperta agli sviluppi e alle innovazioni dell'agricoltura, che guardava certamente all'Italia, ma anche e sempre alle esperienze degli altri Paesi europei. *(Applausi)*.

con la scomparsa di Romualdo Coviello la Basilicata e il Paese intero perdono un uomo di altissima levatura, che ha messo le sue grandissime competenze in campo economico e agrario a servizio della nostra Regione e dell'Italia intera. Ha incarnato ai massimi livelli istituzionali le spinte migliori che hanno animato la tradizione popolare della Democrazia Cristiana. La sua azione politica e amministrativa non ha mai sofferto del difetto dell'improvvisazione dettata dall'urgenza. Ha sempre improntato il suo agire a una visione ampia e lungimirante. Mi lega a lui il periodo della mia formazione giovanile quando, ancora studente, muovevo i primi passi nella politica regionale. Prima ancora ricordo quando, pieno di ammirazione, lo ascoltai intervenire nel metapontino, dove era andato per inaugurare una delle prime sagre della fragola. Oggi la Basilicata detiene il primato in questa filiera e sicuramente un po' è anche merito suo. Ho un vivo ricordo del suo esempio politico con la centralità data proprio all'agricoltura e la ferma volontà di sviluppare e ammodernare la Basilicata proprio a partire dal settore primario. Conservo intatta nei miei ricordi la sua immagine di assessore regionale, quando affrontava i problemi dei nostri agricoltori lucani con decisione e risolutezza. Negli uffici regionali sentono ancora le sue urla quando gli agricoltori si lamentavano che non gli arrivava l'acqua per le colture stagionali e lui alzava il telefono per redarguire i vari enti preposti, il consorzio di bonifica o l'ente di irrigazione. Gli agricoltori per lui erano sacri, eredità ricevuta dal suocero compianto Decio Scardaccione. Mi lega inoltre a Coviello il suo impegno politico e istituzionale per il riscatto e l'emancipazione delle aree più deboli del nostro Paese. Nel 2004, illustrando alcune mozioni sul Mezzogiorno, evidenziava come la strategia politica del Governo per il Sud dovesse essere mirata alla redistribuzione complessiva delle risorse destinate agli squilibri interni, affinché il Mezzogiorno fosse in grado di cogliere le opportunità e di diventare un'area di libero scambio nel Mediterraneo. Anche in sede di riforma in senso federalista dello Stato riteneva che le peculiarità del Sud dovessero essere tenute in debita considerazione per accorciare il forte divario esistente tra le due aree del Paese. Al fine di impedire un ulteriore arretramento del Mezzogiorno proponeva di valorizzare le istituzioni e i soggetti economici meridionali; di destinare una quota maggiore di investimenti pubblici alle infrastrutture e ai sistemi di rete; ponendo nel contempo l'accento sulla qualità dello sviluppo e sul contrasto a ogni forma di illegalità. Da economista aveva ben chiaro il concetto di interdipendenza economica e gli effetti benefici per il Nord degli investimenti effettuati al Sud. Unitamente a ciò, sul piano istituzionale, riteneva che occorresse indirizzarsi sulla strada di un federalismo solidale che, in una sede politica alta e unitaria, si facesse carico di contemperare le esigenze dei diversi territori, nel presupposto che lo sviluppo del Paese non potesse essere scisso da quello del Mezzogiorno. Dunque, è un esempio di cattolico impegnato attivamente nella politica a servizio della gente. Nel suo indimenticabile ricordo, continueremo a lavorare perché le sue intuizioni e i suoi insegnamenti siano un prezioso lascito per tutti i lucani, per tutti gli italiani e per noi parlamentari. Grazie Coviello.

ho l'onore di ricordare in quest'Aula una personalità autorevolissima, importante per la Basilicata, il senatore Romualdo Coviello, che ci ha lasciati qualche giorno fa; una personalità che ha che ha fatto tanto per la nostra Regione e, in un'ottica di unità della Nazione, anche per l'intero Mezzogiorno. prima lei ha ricordato il percorso istituzionale del senatore Romualdo Coviello. Mi piace aggiungere che egli è stato tra i costituenti dell'ente Regione Basilicata,

quale quello di Presidente del Consiglio regionale. Ribadisco anche il fatto che sia stato un eccellentissimo rappresentante parlamentare di questo ramo del Parlamento, per altri circa venti anni, dove ha saputo portare le istanze del suo territorio; quel territorio che annaspava, che era in sofferenza, in difficoltà rispetto al resto del Paese e che doveva recuperare un ritardo che non poteva più essere giustificato. ha saputo coniugare il ruolo istituzionale - per quanto appena detto - e il ruolo politico. Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, ma ne ho sentito parlare, tanto tanto e bene. Mi raccontano che non disdegnava affatto la militanza politica. Diceva prima il collega Pittella che sapeva guardare lontano, ma sapeva anche tenere le orecchie a terra - come si suol dire stare vicino al territorio e alla propria gente, in aggiunta all'impegno anche accademico. Tutto questo lo ha condotto a portare avanti la teoria di uno sviluppo autopropulsivo della nostra Regione, una teoria che ritengo sia attualissima.

lo meritava tutto. Da giovane rappresentante istituzionale della Basilicata, rivolgo il seguente auspicio, intanto a me e a tutta la classe dirigente lucana che si avvia a intraprendere un percorso: mutuare un insegnamento dal senatore Romualdo Coviello, sarebbe quello di portare avanti l'impegno politico e istituzionale con dedizione, con passione e tanto studio, che non guasta mai. Per questo, a nome e per conto del Gruppo del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, giunga ai figli del compianto senatore Romualdo Coviello, ai familiari e a tutti i suoi cari, il nostro sentito, rispettoso, affettuoso e commosso saluto. *(Applausi)*.

di un argomento che sicuramente, in questi giorni, è all'attenzione un po' di tutti i cittadini, e cioè il dibattito sull'alimentazione. Approfitto dell'occasione per salutare e ringraziare, in rappresentanza del Governo, il sottosegretario Centinaio, che su questo argomento, insieme al ministro Patuanelli,

nuova visione dell'alimentazione e di come considerare il rispetto dell'ambiente da qui alle prossime scadenze visionate dalla Commissione europea; Commissione europea ridurre le emissioni in atmosfera, spesso e volentieri dando la colpa agli agricoltori e un po' anche all'alimentazione del nostro Paese; punto che stanno rimettendo in discussione con il nutri-score. Approfitto dell'occasione per

grande qualità della produzione dei nostri agricoltori, a cui va veramente il mio complimento, perché siamo il Paese della biodiversità: in Italia ricordo che abbiamo abbiamo oltre 7.000 specie vegetali commestibili. Non capiamo pertanto come mai con il nutri-score spesso e volentieri i nostri prodotti siano etichettati con il bollino rosso.

con la dieta mediterranea e soprattutto con il *made in Italy*, siamo forse il Paese più longevo al mondo; dico forse perché siamo superati di poco dal dal Giappone che, come longevità, ci supera forse di un anno, e non di più. Se siamo il secondo Paese al mondo per longevità, significa che mangiamo bene, che il *made in Italy* va sicuramente salvaguardato e che il nutri-score non ha assolutamente nulla a che vedere con il nostro sistema alimentare.

perché, la Commissione agricoltura si è dimostrata compatta come non mai; in terzo luogo, perché, se siamo tutti uniti in maniera granitica e lavoriamo tutti in un'unica direzione, forse riusciamo a spuntarla nei confronti della Commissione europea che - voglio ricordare - non più di un mese fa ha autorizzato i cittadini a mangiare i grilli,

che è quella di valorizzare il grande lavoro e la qualità dei prodotti degli agricoltori italiani, che vanno difesi tutti assieme.

Signor Presidente, signor Sottosegretario - non vedo il Ministro - colleghe e colleghi, l'Europa ci chiede sempre e ci chiede ancora, ma toglie - almeno all'Italia - e non dà. Non mi richiamate il PNRR, perché tutti sappiamo che parte di quei soldi li dovremo restituire Ci toglie quando alcuni Paesi dell'Unione europea (Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) adottano il nutri-score: un semaforino rosso con il quale bocciano i nostri prodotti d'eccellenza facenti parte della dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'UNESCO. E poi sicuramente penalizzerà i nostri prodotti con il piano decennale del Farm to fork, che, se non gestito bene e armonizzato con tutti i Paesi europei, ci porterà dei danni, considerando che già l'Italia ha una grande attenzione verso verso la sostenibilità ambientale e la biodiversità, che garantiscono appunto la qualità della produzione *made in Italy*. Se il Farm to fork deve essere, *in primis* deve essere per ogni Paese dell'Unione europea e tutti si devono uniformare a questo programma - purtroppo leggo che non è vincolante - con armonizzazione di mezzi e di tempi, attraverso i piani strategici nazionali. Ma preliminarmente, considerato che ci sarà un calo della produzione anche del 30 per cento, perché sostanzialmente non si andranno a usare tante sostanze - ed è pur giusto così - dobbiamo in qualche modo pretendere che tutti i prodotti che entreranno in Italia dai Paesi terzi, e che verranno a propinarci, non siano trattati con ogni tipo di sostanza da noi vietata, magari pregiudicando anche la nostra ridotta produzione. Sarebbe interessante - ma il Ministro non c'è - sapere com'è andata a finire la rinegoziazione del trattato bicamerale con i Paesi del Nord Africa per quanto riguarda la filiera agrumicola. Ma non ci è dato sapere. Colgo l'occasione come portavoce del nascente Coordinamento produttori ortofrutticoli italiani, che, attraverso me, invita il ministro Patuanelli a tutelare i produttori di questa filiera, danneggiati dalla pandemia, dalle variazioni climatiche e soprattutto dall'aumento delle materie prime, non hanno i soldi e la liquidità per organizzare la prossima campagna produttiva e chiedono a gran voce che nel

entro il 2030 dovremo garantire la protezione di almeno il 30 per cento delle aree rurali e marine europee; trasformare il 10 per cento delle superfici agricole in aree ad alta biodiversità;

È un'occasione storica per cambiare il corso dello sviluppo europeo e per portarlo al passo con i tempi che viviamo, che impongono una transizione di pensiero, prima ancora che energetica o produttiva. Il sistema agroalimentare italiano offre la maggiore garanzia di qualità e salubrità a livello mondiale. Non per nulla, la dieta mediterranea è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO. L'Italia, forte del suo primato, sostiene il sistema di etichettatura nutrinform, rispetto al nutri-score voluto da altri Paesi europei, che hanno una tradizione agricola diversa dalla nostra. L'obiettivo è quello di informare i cittadini europei su ciò che mettono sulle loro tavole. Purtroppo i diversi Stati membri non sembrano mostrare quell'armonia raccomandata dalla strategia europea e, in sede europea, sembra esservi una propensione per il sistema di etichettatura denominato nutri-score, che è stato adottato in Francia nell'ottobre 2017. I motivi di perplessità delle etichette a semaforo sono diversi. Innanzitutto, alcuni esperti hanno fatto notare come l'algoritmo utilizzato per assegnare i colori ai vari prodotti sia poco trasparente. Inoltre, il criterio dei colori è troppo riduttivo e semplicistico, per cui di fatto risulta più un'induzione al consumo, una sorta di strategia di *marketing*, che una vera informazione nutrizionale su base scientifica. Infine, ma non per ultimo, ciò che l'Italia contesta a questo sistema è che nessun cibo è buono o cattivo di per sé, ma deve essere valutato in base al suo apporto quotidiano di energia, sali, zuccheri e proteine, nell'ambito dell'intera dieta del consumatore. In base a questo sistema - ad esempio - ci troviamo di fronte al paradosso per cui una bevanda gassata o con edulcoranti, oppure la carne sintetica, appaiono più sani di un cucchiaio di olio d'oliva o di un pezzo di parmigiano. È evidente che c'è qualcosa che non va in questo sistema. L'Italia ha proposto un sistema alternativo a batteria denominato nutrinform, che parte da un criterio completamente diverso dal nutri-score, dal momento che valuta il ruolo strategico del singolo prodotto all'interno della dieta. Una buona cultura alimentare si basa sull'educazione e sulle scelte consapevoli dei consumatori, con una dieta varia che non escluda alcun alimento, ma ne consenta il consumo secondo frequenze e porzioni adeguate. Il rischio principale di un sistema fuorviante come il nutri-score è di penalizzare fortemente sui mercati i prodotti d'eccellenza del nostro *made in Italy*. Del resto, le attività di pressione per fare concorrenza all'agroalimentare italiano non sono certo una novità. Importante sarebbe spingere la Commissione a realizzare massicce campagne informative: non basta sapere cosa si compra, ma anche le quantità da consumare. Occorre fare un passo in più: un cibo sano innanzi tutto, quello che viene prodotto con pratiche sostenibili non impattanti sugli ecosistemi. L'agricoltura biologica in questo è la migliore garanzia della salubrità degli alimenti; i consumatori devono essere consapevoli se nel cibo siano presenti o meno residui di pesticidi o di altri contaminanti. Tra l'altro, tutto questo avrebbe un potente effetto di prevenzione sanitaria che ridurrebbe i costi del nostro bilancio sanitario. Per questi motivi, nella mozione firmata insieme ad altri colleghi della Commissione agricoltura, abbiamo chiesto vari impegni al Governo. Auspico vivamente che il Governo voglia raccogliere tali impegni e che l'Italia in generale muova passi concreti e decisivi verso un'agricoltura sostenibile, dignitosa per gli agricoltori - guardiani del nostro paesaggio e dell'ambiente - e attenta ai bisogni dei cittadini.

vide la partecipazione di un grande uomo, un grande imprenditore, una grande persona, un esempio di forza di volontà, altruismo e responsabilità. Mi riferisco a Ennio Doris, e, visto che è mancato recentemente, direi anche di rivolgergli un applauso. ci raccontò di un'unica penisola al mondo stretta da Nord a Sud dentro a un mare buono, buoni dei nostri mari incontrano l'aria fresca dei monti, creando una situazione unica al mondo. Da lì nascono alcuni prodotti quali - ad esempio - il prosciutto crudo San Daniele, figlio della bora e delle Dolomiti; il crudo di Parma, figlio delle Alpi Apuane e del Mediterraneo; la pasta più buona al mondo, quella di Gragnano, che si crea dove si incontra l'aria fresca di Castellammare di Stabia

del mondo. Come ricordava prima il presidente della Commissione agricoltura Vallardi, in Italia abbiamo 7.000 specie vegetali mangiabili, ricordando che il Brasile è secondo con 3.300 vegetali. Abbiamo 58.000 specie animali, 42.000 di terra e aria, 10.500 di acqua salata e 5.500 di acqua dolce. Siamo il secondo Paese al mondo per le specie animali. Abbiamo 1.200 vitigni autoctoni, la Francia che è seconda ne ha 222; 533 cultivar di olive (la Spagna, seconda, ne ha 70). Abbiamo un'enorme ricchezza di biodiversità trasformata nel nostro patrimonio agroalimentare. Faccio un esempio. È fuorviante che con il nutri-score si faccia riferimento a 100 grammi di prodotto, quando la diversità di un pasto dispiega i suoi benefici grazie a una moltitudine di elementi nutritivi. Abbiamo mille esempi a livello nazionale: se 100 grammi di carne vengono indicati dal nutri-score come sostanza pericolosa o cancerogena, è associata una varietà, una moltitudine di prodotti vegetali che hanno elementi nutritivi molto importanti, benefici che derivano dalla ricchezza del piatto, e non una ricchezza nutritiva di 100 grammi. grammi. Il nostro compito, quindi, è educare a una cultura del consumo sano, come lo è la nostra dieta mediterranea, che è patrimonio UNESCO. Abbiamo un patrimonio storico fatto di culture che hanno trasformato la biodiversità italiana in migliaia di piatti e portate.

quindi ai ringraziamenti al presidente Vallardi e a tutta la Commissione, che unitariamente ha sottoscritto questa mozione. L'unione fa la forza, e lo abbiamo visto anche nella battaglia che stiamo portando avanti con il Prosek, quale siamo uniti soprattutto per questioni legate al nostro Paese. In ambito agroalimentare, a difesa del *made in Italy*, sicuramente raggiungeremo obiettivi importanti contrastando la cultura dell'omologazione. la mozione appena illustrata pone una questione di non secondaria importanza soprattutto per il nostro interesse nazionale, che racchiude gli interessi della miriade di piccole e medie aziende nostrane, se non la loro stessa esistenza sul mercato. È soprattutto per questo che il nostro Governo deve farsi valere sul piano europeo con voce autorevole e assertiva, ma non soltanto per questo. I due concetti che convergono sono quelli della Farm to fork e del nutri-score. Nel primo va ravvisata una precisa strategia che tocca molti aspetti dell'intera filiera agroalimentare, che parte dai campi, passa dal criterio da adottare per l'etichettatura - criterio che non va assolutamente sottovalutato - e giunge fino alla forchetta, appunto, che - mi si perdoni la digressione - è un oggetto che il raffinato artigiano italiano di matrice umanistica ha donato al mondo intero. Sui due modelli da adottare per l'etichettatura, che attualmente si contrappongono e animano il dibattito in sede europea, cioè sul nutri-score da una parte e dall'altra quello della nutrinform battery, non è indifferente l'opzione per l'uno o per l'altra, risultando il primo fuorviante e penalizzante per la produzione nostrana e per un settore economico così importante. Ma non è soltanto questa la criticità che si annida nel nutri-score. Infatti, il nutri-score che tanto piace ai Paesi del Nord risulta essere parziale e fuorviante per il consumatore finale, perché nella valutazione della bontà di un alimento o di una bevanda prende in considerazione una soglia minima arbitraria, rispettivamente una quantità di 100 grammi per gli alimenti e 100 milligrammi per le bevande. Il nutri-score, quindi, non tiene conto dell'assicurazione giornaliera di alimenti e bevande, non tiene conto della porzione. La nutrinform battery, cioè la proposta italiana, invece non si basa sul mero aspetto nutrizionale del singolo alimento o della singola bevanda. È un criterio che li inserisce in una dieta complessiva varia e bilanciata; va cioè a recuperare i principi basilari della dieta mediterranea, che - come ho avuto già modo di dire in questa stessa sede - ha una riconosciuta capacità di prevenire le malattie cronico-degenerative; una dieta che un sapere secolare rispettoso delle stagionalità e dell'effettivo fabbisogno nutrizionale ha delle conseguenze salutari nel breve, ma anche nel lungo termine. questo, la posizione dell'Unione europea sull'impiego dell'etichettatura non è ancora definita; attualmente ogni Stato membro è libero di adottare uno schema di etichettatura applicato volontariamente dagli operatori del settore alimentare. che una faccenda così delicata non può essere affidata solo alla buona coscienza dei produttori *(Applausi)*, tanto più perché i nostri prodotti sono minacciati da due formidabili insidie: dalle agromafie, che tendono a insediarsi in ogni segmento della produzione e distribuzione, e dall'*italian sounding,* oltre che dalla contraffazione, che rappresentano un grande danno per l'economia italiana, implicando un volume d'affari di circa 500 miliardi di euro annuali. Ricordiamoci che, su tre prodotti di marchio italiano venduti nel mondo, ben due sono in realtà contraffatti. Ben vengano quindi iniziative come quella promossa dalla *start up* napoletana Autentico, che ha creato un'*app* che, scandendo il codice a barre, permette di sapere se un prodotto è un vero *made in Italy.* Il nutri-score, così come è concepito, penalizza le eccellenze agroalimentari nostrane, è di facile fruizione e molto intuitivo, ma - come ho cercato di argomentare - è ingannevole per il consumatore e penalizzante per la nostra economia

cercando di dare un taglio più sanitario al mio contributo, vorrei ricordare come l'Italia abbia dei dati molto preoccupanti sull'obesità infantile. Una recente indagine

L'obesità dei primi anni di vita è alla base di una serie di patologie che si svilupperanno nel corso della vita, con una notevole incidenza sulla spesa sanitaria e una popolazione meno protetta dalle malattie. Diete ricche di carboidrati raffinati, grassi e zuccheri sono la causa principale dell'obesità, così come di altre disfunzioni: pensiamo all'esplosione delle intolleranze e delle allergie collegate all'assunzione sistematica di alimenti e bevande che vedono una forte presenza di elementi chimici per la loro produzione. Pensiamo altresì all'esplosione di malattie metaboliche come il diabete che, con le loro complicanze, sono devastanti per l'organismo umano. Anche per questa ragione, signor Presidente, gli impegni posti dal Parlamento europeo col programma Farm to fork sono di grande importanza. Lo sviluppo di produzioni biologiche, lo stop ai pesticidi, il contrasto agli allevamenti intensivi, l'accorciamento delle filiere sono tutti elementi che vanno in questa direzione. Come medico lo reputo uno degli elementi di maggior pregio dell'impegno che l'Europa si è data come cornice di una maggiore sostenibilità ambientale dell'intero settore. Non possiamo, infatti, non vedere quanto l'industria alimentare rappresenti una delle principali forme di inquinamento e, quindi, una minaccia per gli equilibri del pianeta. Non possiamo poi dimenticare che gli allevamenti intensivi - ad esempio - col costante disboscamento di parti del pianeta, abbiano rotto una serie di equilibri che sono alla base delle ultime epidemie, compresa naturalmente quella del Covid-19 che purtroppo stiamo vivendo. È chiaro È chiaro che questi obiettivi devono essere raggiunti con un percorso graduale e non solo nel tessuto industriale. Dobbiamo scongiurare il rischio che la strategia Farm to fork riduca il nostro potenziale produttivo, aprendo le porte a importazioni che per nulla contribuirebbero agli obiettivi che si pone. Dobbiamo altresì scongiurare che questa transizione venga pagata di propria tasca dai cittadini. Così come vanno ascoltate con molta attenzione le questioni di chi si pone il tema di un altro tipo di sostenibilità, ossia quanto gli attuali modelli siano efficaci rispetto a una domanda alimentare chiamata a sfamare un pianeta in costante crescita demografica. Allora l'unica strada che abbiamo è quella di puntare - da un lato - sullo sviluppo e sulla ricerca per conciliare tutte queste esigenze e - dall'altro su una sana cultura dell'alimentazione, ossia su una sempre maggiore consapevolezza da parte dei cittadini del loro rapporto con il cibo. Anche su questo, signor Presidente, l'Unione europea non deve commettere un errore, ma deve fare un salto di qualità sul discorso dell'etichettatura dei prodotti. Bisogna passare dal modello nutri-score, che ragiona in maniera assolutistica su un singolo cibo, a quello nutrinform, che illustra la giusta quantità di cibo assumibile quotidianamente. Questo perché la salute, come dicevo prima, passa dalla costruzione di diete equilibrate e non da questo o quel bene di consumo. Dobbiamo impegnarci per formaggi e carne di qualità, in cui vengano usati sempre meno additivi, esattamente come nel caso dei biscotti che, nel giro di un paio di anni, hanno rimosso l'uso dell'olio di palma e di grassi idrogenati. Poi, chiaramente, questi prodotti dovranno essere bilanciati all'interno di una dieta. Ricordiamoci che un'alimentazione sana, corretta e bilanciata, insieme a una costante attività fisica, rappresenta il pilastro fondamentale della prevenzione primaria, cioè quella strategia di politiche sanitarie principali per ridurre l'incidenza delle malattie metaboliche e cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di morte e disabilità grave in tutto il mondo occidentale. Pertanto, la battaglia italiana in sede europea non è solo giusta per la difesa delle nostre imprese, ma

la volontà di tutte le forze politiche, nessuna esclusa, di porre un argine non solo ideologico, ma anche scientifico

oggi è finalmente patrimonio di tutta l'Assemblea e le forze politiche quanto sia assolutamente anti-italiano e contro i prodotti italiani questo tentativo

delle Nazioni europee per renderci conto di come questo uso un po' farfallino della salute venga strumentalizzato proprio nel momento in cui mancano gli argomenti e la salute è l'unico collante che consente alle forze politiche di mantenere di mantenere il proprio *status.* Ora, concentrandoci sulla strategia Farm to fork, avremmo non solo una critica diretta ma anche qualcosa da dire rispetto a certe attestazioni più ideologiche che utili, come quelle che il documento Farm to fork sancisce. Abbiamo denunciato dal primo momento il porre dei vincoli all'Europa senza guardare a ciò che fanno Nazioni molto più inquinanti e meno attente alla

che è un tutt'uno con noi e non qualcosa di terzo rispetto a noi, dobbiamo interrogarci su come riuscire poi a sfamare una popolazione del mondo che è in assoluta crescita. Rischiamo altrimenti altrimenti di scrivere bellissime pagine di antologia e filosofia e poi non essere in grado di far sì che tutti,

europea è riuscita a fare negli ultimi anni. Parlo di questo perché mi sembra evidente che ci sia stata più ideologia che innovazione nel documento al nostro

onori della cronaca perché in questo si è letto una forte penalizzazione del comparto agricolo, cosa che tra l'altro si tradurrebbe nell'immediato, ma semplicemente perché questo strumento penalizza tutta la filiera italiana, dall'agricoltura a chi fa le esportazioni, dalle case di trasformazione a chi si occupa di mantenere il territorio.

e sono le stesse persone che oggi ci stanno aiutando a manifestare con chiarezza l'antiscientificità di queste operazioni, ma anche la soluzione. È forse questo il primo campanello che dovrebbe suonare, quello cioè di dire che abbiamo oggi in Italia delle professionalità tali che non solo ci consentono di avvertire per primi il pericolo, ma ci consentono addirittura con l'elaborazione e con l'aiuto di tante imprese private di elaborare la risposta a questi problemi. Il nutrinform battery è infatti la risposta a questi problemi ed è frutto della grande partecipazione di tutti i soggetti politici, di tutti i soggetti tecnici e anche di soggetti privati che si sono messi a disposizione; Federalimentare, l'Università della Luiss, tutte persone che hanno costruito la nostra posizione contro il nutri-score. Se fosse stata una posizione meramente politica, di contrapposizione fra Stati e fra Nazioni, con molta probabilità gli interessi che hanno dominato fino ad oggi quelle Nazioni, nelle quali il nutri-score è fiorito, ci avrebbero massacrati sotto il profilo delle evidenze scientifiche. Oggi invece dobbiamo ringraziare il grande lavoro tecnico che abbiamo fatto nei Ministeri. Ringrazio il sottosegretario Centinaio per ringraziare in questo caso tutta la struttura. È palese, qualcuno deve avere l'onestà anche intellettuale di dirvi le cose quando non funzionano, ma di dirvi che noi, Nazione Italia, indipendentemente da chi oggi è al Governo, possiamo contare su delle professionalità assolutamente valide. A queste però vanno aggiunte altre professionalità che ci consentono uno *step* superiore, vale a dire aumentare l'innovazione in agricoltura, per tornare alle rese del 1984, per citare un esempio classico

l'agricoltura al livello che merita, cioè a un settore primario non solo nel nome, ma anche nella considerazione generale. Anche perché l'agricoltura pulita e sostenibile è quella che i nostri agricoltori fanno già, signori.

sul fronte agricolo: si taglia e si pretende da tutti la stessa diminuzione, ad esempio dell'uso dei fitofarmaci, quando sappiamo tutti che l'Italia è il sesto Paese al mondo per l'utilizzo graduale di fitofarmaci. Non conosco un solo agricoltore che che avveleni il proprio terreno nella piena consapevolezza del fatto che l'anno dopo deve tornare a lavorarlo: nessuno si suicida in agricoltura. però sfide ancor più globali, come il cambiamento climatico, che devono consentire ai nostri agricoltori di avere quegli strumenti, anche chimici, purtroppo, per una quota parte, fino a quando non troveremo un sistema naturale che sostituisca il sistema chimico. Come quando è malato un corpo umano, anche una pianta, anche un

(della quale ringrazio tutti i colleghi, perché anche questa volta siamo arrivati a un atto completamente condiviso e costruito insieme), di un tema per noi sostanziale. Sono quasi due anni che parliamo di quanto sia importante - e in quest'Aula lo abbiamo ripetuto tante volte - il settore dell'agroalimentare; ce ne siamo accorti soprattutto in questa pandemia, nella quale mai un giorno è mancato un alimento sui banchi dei nostri supermercati e durante la quale si è avuto maggior tempo per conoscere i nostri prodotti. Alcune ricerche in questo senso dimostrano quanto, soprattutto nel primo momento della pandemia, si sia tornati a guardare con accuratezza e con interesse a ciò che si mangia.

È determinante conoscere e costruire un regime alimentare e uno stile di vita sano e, quindi, costruire la nostra dieta in modo che possa corrispondere anche al nostro benessere. Questo ci dice che costruire un'etichetta su un prodotto alimentare diventa sostanziale, fondamentale. È per questo che siamo contro un sistema, quello del nutri-score, dà informazioni come se dovessimo mangiare solo e soltanto un determinato alimento, solo e soltanto un determinato nutriente, tirandolo fuori da un contesto che è quello, invece, di un regime alimentare bilanciato e vario, che tutti i nutrizionisti e anche i medici ci dicono di seguire. Non viene inserito, nel nutri-score, questo elemento fondamentale di bilanciamento della dieta e di varietà della stessa, facendo prima di tutto un danno a chi consuma quel determinato alimento. È impensabile che si mangi soltanto una cosa, mentre l'etichettatura del nutri-score fa intendere esattamente quello, con questi colori e queste lettere, che riportano soltanto la constatazione e la considerazione di un alimento, che può fare più o meno male: come se dovessimo nutrirci esclusivamente di carote o di finocchi e, da un'altra parte, soltanto di dolci,

l'alimento che va a comprare, lo inserisca nel suo regime alimentare, nella sua dieta, in modo da poter poi seguire uno stile di vita sano. Il tema non è, quindi, guardare soltanto a un singolo nutriente e a un singolo alimento, ma di considerarlo: l'ho già detto, ma questo è un punto fondamentale per capire la dannosità del nutri-score e, invece, le potenzialità del nutrinform battery, che è il sistema che, secondo noi, deve essere all'interno delle nostre abitudini alimentari. Il troppo stroppia: questo porta al nutri-score, che secondo noi è un metodo sbagliato. La nostra dieta mediterranea ci insegna molto bene che la varietà, con ogni singolo alimento che deve essere inserito all'interno di essa, è il massimo per quanto riguarda la nutrizione. Questo comporta anche la tutela dei nostri presidi alimentari e dei nostri prodotti di alta qualità. Sicuramente l'Italia ne può vantare tantissimi, ma, non è soltanto una questione italiana. Ciascun Paese ha degli alimenti di ottima qualità, che dovrebbe avere interesse a garantire, dei presidi che dovrebbe avere interesse a garantire. Non si capisce perché, quindi, in Europa questo messaggio non passi. Parliamo del nostro vino, del nostro olio, dei nostri formaggi, dei nostri salumi delle nostre carni. Alimenti di altissima qualità, che sono frutto anche di investimenti importanti fatti in questo ambito.

Presidenza, facciamo pervenire al Governo è l'invito a difendere prima di tutto la cultura del mangiar bene, la cultura del cibo sano e, soprattutto, di uno stile di vita sano. obiettivo, secondo noi, è perseguibile solo e soltanto con il nutrinform battery. E speriamo che l'Europa si renda conto che, in questo modo, ogni Paese riuscirà a preservare al meglio anche i propri presidi di qualità alimentare.

Signor Presidente, una novità? Direi proprio di no: il nutri-score è quel sistema di etichettatura a semaforo proposto dalla Francia che assegna un colore, dunque un via libera o meno, ad ogni alimento in base al livello di zuccheri, grassi e sali calcolati sulla base di riferimento di 100 grammi di prodotto. Intuitivamente, quindi, cibi verdi, ossia col semaforo verde, sono da preferire rispetto a quelli rossi. Capite bene che cibi di grande importanza per il nostro patrimonio agroalimentare, come l'olio d'oliva, il parmigiano reggiano o anche il prosciutto di Parma, diventerebbero alimenti sconsigliati dal nutri-score. Perché non è una novità? Perché questo tira e molla politico sul comparto alimentare è diventato ormai una consuetudine fastidiosa che in Europa ritorna puntuale andare a infierire in maniera importante su quei tratti caratteristici distintivi e rappresentativi del valore aggiunto di un'economia, quella agroalimentare italiana, vuol dire in realtà poterla controllare e acquisire le sue quote di mercato, quindi è una vera e propria battaglia economica. Chi per morfologia, cultura e clima deve rifarsi a colture di carattere intensivo e Nazioni che hanno evidenti interessi di concorrenza rispetto alla qualità delle nostre produzioni alimentari è chiaro che iniziano a guardare al settore primario come un ulteriore elemento che sposta l'ago del potere. Dopo tutto, se l'industrializzazione e l'economia conoscono andamenti sinusoidali legati ai mercati, alle tecnologie, all'evoluzione della società e altri mille fattori, è pur vero che, ancorché involutivo nella propria modalità di vita, l'essere umano non può prescindere dall'alimentazione: sono ormai anni che assistiamo a continui attacchi al nostro *made in Italy* e alla nostra dieta: dagli impedimenti del diritto doganale nel regolamento n. 1169 del 2011, dove basta la trasformazione e non l'origine della materia prima per definire un *made in*, all'annosa questione delle colture OGM di bassa qualità, spinti comunque sempre - guarda caso - dalle *lobby* tedesche. Oggi l'evoluzione della legislazione europea porta ai fenomeni dell'etichettatura a semaforo e al *cancer plan*. Il primo, ovvero il nutri-score, non tiene conto dell'integrazione degli elementi della dieta: abbiamo detto che si occupa esclusivamente di fare la lista dei buoni e dei cattivi, senza dare nessun peso a una dieta equilibrata. ne approfitta, per esempio, per inserire il vino nella lista dei prodotti a impatto cancerogeno (ovviamente, un basso consumo di vino non è cancerogeno). Due modalità parallele che, per loro stessa natura, non si incontreranno anche se parlano della stessa cosa, ovvero dell'alimentazione e della salute. Peraltro, così facendo si va a penalizzare proprio chi, come l'Italia, è sempre stato portabandiera della dieta mediterranea, suoi benefici e dell'uso responsabile, sano e integrato degli alcolici come il vino che, a parte casi sporadici per i quali andrebbe aperta un'altra finestra di discussione, ha fatto della salubrità, della correttezza alimentare come strumento di benessere e longevità e della ricerca multiculturale il suo basamento economico e culturale. Vorrei aprire una piccola finestra sulla salute e vorrei anche capire più in là, quando sarà possibile, quale sia la reale posizione del ministro Speranza, visto che Walter Ricciardi, consigliere del ministro Speranza, si è chiaramente schierato a favore del nutri-score. Questo andrebbe a cozzare fortemente con gli interessi del nostro Paese, a meno che non si sia deciso che il Governo prenda un'altra strada. Qui la sanità non c'entra; c'entra l'economia, perché la *ratio* del nostro sistema a batteria è proprio questa: coniugare la qualità, le proprietà organolettiche dei cibi e mettere tutto in un'integrazione con una dieta sana come quella mediterranea, che - dovremmo spiegarlo ai signori della Commissione europea - aiuta a prevenire il cancro e non lo induce.

è una grande fesseria scientifica dire che il nutri-score fa bene alla salute. In un periodo in cui l'anti-scienza fa paura, bisognerebbe evitare di portarla nel settore agroalimentare con delle teorie del tutto folli come quelle secondo cui mettere un semaforo agli alimenti potrebbe dare una dieta equilibrata. quindi che, come in Commissione agricoltura abbiamo sottoscritto in maniera unanime questa mozione, anche questo Parlamento esprima un no unanime al nutri-score e questo dia la forza al nostro Governo di andare a far valere questa posizione controversa nelle sedi europee e dire no al nutri-score sia per questioni economiche, che per questione di salute pubblica.

perché hanno portato all'attenzione dell'Aula un argomento molto interessante. Il *green deal*, con l'intento di ridurre le emissioni di gas serra entro il 2050, attraverso una transizione ecosostenibile dei sistemi di produzione e di lavorazione, ha due strumenti particolari di attuazione: una strategia che è stata definita Farm to fork e la strategia sulla biodiversità. Queste due strategie hanno obiettivi ambiziosi da raggiungere entro il 2030. Ricordo, tra gli altri: un incremento del 25 per cento delle superfici coltivate a biologico, una riduzione del 50 per cento dell'uso dei fitofarmaci, una maggiore efficienza dell'uso dei nutrienti azoto e fosforo, che porterà a una riduzione dell'utilizzo dei fertilizzanti stimata nell'ordine del 50 Attenzione, colleghi, però, perché le parole sono scritte bene: non è un aumento del 25 per cento dell'agricoltura bio, ma bisogna arrivare ad avere almeno il 25 per cento dei terreni coltivati a bio in Europa. Piccola, ma non banale questione. Altro argomento, signor Sottosegretario: si calcola sul totale delle superfici coltivate dell'Unione europea o di ogni singolo Stato aderente? L'Italia, per esempio, è già *leader*, con quasi il 20 per cento delle superfici coltivate a bio. Quindi l'Italia può arrivare al 25 per cento attraverso queste due strategie, ma in altri Stati dell'Unione si parte quasi da zero (pensiamo all'Ungheria, al Nord Europa, alla Polonia, alla Croazia). obiettivi condivisibili, sia chiaro, colleghi, ma manca una valutazione effettiva dell'impatto globale di questi obiettivi sul settore agroalimentare. Sono obiettivi che rischiano di ridurre la competitività dell'agricoltura europea, in particolar modo dell'agricoltura italiana. Non solo il Dipartimento federale dell'agricoltura americano ha stabilito, ma anche la più autorevole autorità del settore, l'università di Wageningen, ha accertato che ci sarà una sensibile riduzione delle produzioni agroalimentari (dal 7 al 12 per cento in meno), che i prezzi al consumo potrebbero aumentare nell'ordine del 17 un aumento delle importazioni da Paesi terzi che non rispettano queste regole e questa normativa. Prima di andare avanti, signor Sottosegretario, serve una preventiva e preliminare valutazione dell'impatto di tali norme. a livello europeo, battetevi con forza, perché è veramente a rischio il nostro comparto agroalimentare. Accanto a queste strategie si inserisce anche il tema dell'etichettatura nutrizionale, che avete definito prima nutri-score. Una piccola autocritica, signor Sottosegretario: è dal 2017 che in Europa stanno parlando di questo argomento. Non lo ascrivo alla sua responsabilità, ma

che si può. Il nutri-score non va assolutamente bene, punisce in maniera anonima - come ha detto il collega De Carlo, che ringrazio - con un taglio verticale tutte le produzioni di eccellenza del nostro Paese, che non sono solo le DOP e le IGP, come il presidente Vallardi ha ricordato molto opportunamente prima.

L'Italia è un esempio in Europa per quanto riguarda le produzioni agricole. Signor Sottosegretario,battete forte i pugni sul tavolo; facciamo capire all'intellighenzia europea che su queste cose non si può scherzare prima di andare avanti con etichette a colori. Ieri mi pare sia stato detto che vogliono mettere il colore nero sul vino. Noi siamo contro l'abuso, non contro l'uso: un sano bicchiere di vino fa bene a tutti. È contro l'abuso che bisogna andare. Non facciamo ideologie su queste cose. Credo che la nostra agricoltura abbia bisogno di un sostegno convinto da tutto il Parlamento.

Signor Presidente, colleghi senatori, rinnovo i dubbi e sollecito gli interrogativi meritevoli di interesse come chi vuole il nutri-score e chi sta strutturando il Farm to fork. Se ci sono politici, ma soprattutto i nostri produttori e le filiere, che muovono molti dubbi, non capisco perché ci siano associazioni che agiscono come *lobby* che invece sono a favore di questo meccanismo subdolo, anche facile da intendere, ma molto vigliacco. È un metodo che paragona la coca cola all'olio di oliva perché sono due liquidi: come se paragonassi uno squalo a un pesciolino rosso perché sono due pesci. *(Applausi)*. È quindi un metodo contro le eccellenze, su una richiesta già ben confezionata e condizionata, ed è fastidioso che, tra le associazioni che fanno parte di Euroconsumers, ci sia anche l'italiana Altroconsumo a favore del nutri-score, con 377.000 iscritti, i quali penso non sappiano che questa fa parte di un *network* internazionale, che il BEUC a cui è iscritto non accetta, fatturando anche 200 milioni l'anno e pare essere indagato anche nei *Panama* *paper*. Oltre a loro, ci sono anche dei quotidiani *on line* sempre a loro legati; quindi, a pensar male è peccato, ma spesso si indovina, come diceva qualcuno. E poi, ci sono ricchi facoltosi che spingono per le bistecche artificiali per poi produrle in bioreattori consumando non solo energia ma anche acqua. soprattutto un fatto: se L'Italia non accetta il nutri-score ne ha anche un'oggettiva ragione, perché la nostra dieta, patrimonio dell'UNESCO, permette una longevità più alta in Europa, una migliore aspettativa di vita - la Germania, ad esempio, è diciassettesima - e il più basso indice di

la difesa della dieta mediterranea, ciò che facciamo nella nostra Commissione, e ringrazio tutti i membri della Commissione agricoltura, a cominciare dal nostro presidente Vallardi, perché noi difendiamo le oltre 1,5 milioni di aziende che ci permettono il 15 per cento del PIL in Italia, con oltre 500 miliardi di fatturato. Insieme al Governo abbiamo fatto anche abbastanza; qualche risultato l'abbiamo ottenuto: la difesa dell'aceto balsamico, della filiera del latte; abbiamo abbassato le accise sulla birra, istituito un fondo per la

gastronomiche, 500.000 euro per le piante aromatiche, 25 milioni per la promozione del vino. Abbiamo difeso il Prosecco dal Prošek e l'etichetta del Chianti italiano abbiamo messo due milioni per la distribuzione delle derrate alimentari, abbiamo voluto l'albo degli agromeccanici e abbiamo anche voluto un fondo di cinque milioni per l'acquisto di macchinari e *software* per l'Agricoltura 4.0. Questo lo facciamo perché ci mettiamo la faccia, e lo facciamo con il sottosegretario Gian Marco Centinaio, persona preparata; quindi, questo è anche il nostro compito di essere al Governo. Il cibo è narratore dell'Italia e se non lo difendiamo perderemo odori e sapori che ci hanno fatto crescere in salute. Il Farm to fork, ovvero dalla fattoria alla tavola, è auspicabile se è dalle fattorie italiane alle tavole di tutto il mondo e non il contrario.

importare frutta e verdura, praticamente la dieta mediterranea. Una maggiore richiesta comporterebbe un maggior costo, una maggiore scarsità di prodotti e un inquinamento della dieta mediterranea e questo è quanto rischiamo

se viene intaccata la nostra dieta mediterranea, sinonimo di buona crescita e salute.

diventano modello di un sistema produttivo più sostenibile, in grado di produrre cibo sano e di qualità per i consumatori europei, garantendo un adeguato guadagno e una maggiore competitività ai produttori. Il documento mira a conseguire gli obiettivi della sostenibilità e del contrasto ai cambiamenti climatici fissati nel *green deal* avviato dalla Commissione europea. Nella mozione presentata dai componenti della 9a Commissione (agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato si condivide la volontà dell'Europa di rendere il sistema agroalimentare ancora più ecocompatibile, senza dimenticare la necessità di riconoscere e compensare i comportamenti virtuosi e guardando sempre all'obiettivo imprescindibile della sostenibilità economica delle imprese, senza la quale non è possibile raggiungere quelle ambientale e sociale. Il percorso segnato dalla strategia Farm to fork dovrà essere incluso anche nelle scelte strategiche del Piano nazionale della futura PAC, la politica agricola europea, prevedendo azioni ed incentivi concreti alle aziende impegnate nell'obiettivo di un sistema produttivo ancora più sano, equo e rispettoso dell'ambiente, al fine di dimezzare il quantitativo di pesticidi chimici entro il 2030. L'eccesso di additivi chimici nell'ambiente è una delle principali cause di contaminazione dell'aria, del suolo e dell'acqua, ha un impatto negativo sulla biodiversità e sul clima, nonché sulla salute umana. L'agricoltura biologica è la pratica che deve essere ulteriormente sviluppata affinché il 25 per cento del totale dei terreni agricoli sia dedicato al biologico entro il 2030. Al fine di aumentare la quota di terreni coltivati secondo pratiche biologiche, è necessario un ulteriore sviluppo lungo tutte le fasi della catena di approvvigionamento e predisporre adeguati incentivi economici per incoraggiare la produzione locale e i canali di distribuzione brevi che consentirebbero agli agricoltori di beneficiare appieno del valore aggiunto dei prodotti biologici, garantendo all'ecosistema il 30 per cento in più di biodiversità rispetto ai terreni coltivati convenzionalmente. Altri obiettivi del piano Farm to fork puntano a migliorare l'informazione ai consumatori attraverso un nuovo sistema di etichettatura europeo degli alimenti e per tale ragione esprimo preoccupazioni sugli ostacoli posti al modello italiano, il nutrinform battery, che colloca le le proprietà nutrizionali di un prodotto in un quadro complessivo di fabbisogno giornaliero, promuovendo in questo modo cibi sani come quelli della dieta mediterranea rispetto a quelli sintetici o processati industrialmente. Occorre quindi che il Governo dispieghi ogni sforzo perché l'Unione europea si doti di un sistema equo e imparziale, che conferisca giudizi scientifici oggettivi rispetto ai valori nutrizionali degli alimenti e che tuteli la salute senza penalizzare le filiere produttive. Allo stesso modo, serve il massimo impegno per impedire qualsiasi forma di discriminazione compiuta ai danni delle eccellenze agroalimentari del nostro Paese che evitino penalizzazioni nell'assegnazione dei fondi europei per la promozione di alimenti, considerando l'alta qualità nutrizionale e l'attenzione verso la sostenibilità ambientale e la biodiversità che le produzioni italiane garantiscono attraverso il delicato connubio tra antica tradizione e innovazione tecnologica. ad esempio, il Parlamento di Strasburgo sarà chiamato a votare il *report* redatto dalla Commissione speciale sulla lotta contro il cancro. Tra queste, c'è anche quella di dotare le bottiglie di vino di un bollino nero, che è una sorta di anticipazione dello scriteriato modo di etichettatura dei prodotti previsto dal nutri-score, il sistema al semaforo prodotto dalla Francia sin dal 2017, che rischia di boicottare alimenti sani del nostro Paese come ad esempio l'olio extravergine d'oliva, il parmigiano, il prosciutto e avendo ovviamente un impatto disastroso sull'intero settore agroalimentare. possibile, colleghi, a questo punto, procrastinare la diffusione di un metodo produttivo compatibile ed in linea con l'approccio agroecologico. Oggi è il giorno in cui l'Italia deve far valere i propri diritti ed acquisire il ruolo guida che le compete nel settore agroalimentare a garanzia della salute dei cittadini, della stabilità economica di migliaia di imprese impegnate nell'agricoltura.

tra chi ritiene che il nutri-score è un progetto fallimentare e tutto il resto, quindi i fautori e gli ideatori del nutri-score.

battaglia europea dell'Italia contro la Francia o contro tutto il resto d'Europa. Vi chiedo semplicemente questo perché diventerebbe una battaglia fallimentare, che andremo a perdere

a mantenere la posizione determinata già assunta in ambito europeo con particolare riferimento alle procedure di attuazione degli interventi del programma di azione, i quali dovrebbero essere preceduti da valutazioni d'impatto approfondite, al fine di garantire la sostenibilità degli interventi stessi, tenuto conto dell'esigenza di individuare i criteri di calcolo e i riferimenti temporali a partire dai quali misurare il conseguimento di ciascun obiettivo; 2) a continuare

il sistema agroalimentare è causa e vittima del cambiamento climatico: causa non solo del 7 per cento delle emissioni inquinanti come sostiene l'ISPRA, ma del 18 per cento se si includono tutte le attività connesse all'attività agricola (dalla produzione dei materiali impiegati, ai consumi energetici e idrici, come ha specificato la FAO). Gli allevamenti intensivi, il disboscamento per il pascolo e l'emissione di metano sono tra le principali cause dei cambiamenti climatici. vittima se si considerano i sempre maggiori danni alla produzione per l'eccessiva siccità o le forte alluvioni, per non parlare - poi - di viaria e peste suina, tutte epidemie legate alla rottura degli equilibri naturali per inseguire il mantra della produzione a tutti i costi. È con grave ritardo che l'Unione europea sta cambiando impostazione sulla politica agricola; per troppo tempo è andata nella direzione sbagliata, favorendo le grandi imprese industrializzate e gli allevamenti intensivi. È ora che le gigantesche sovvenzioni non vadano più soltanto ai più grandi, ma che finalmente una parte vada anche ai più virtuosi, tra cui quell'agricoltura di montagna troppo spesso penalizzata dalle scelte europee. Qualcosa si sta smuovendo, ma non è ancora abbastanza. L'agricoltura di montagna, con le sue produzioni di nicchia, svolge da sempre una funzione preziosa di presidio del territorio, disincentivo allo spopolamento e contrasto al dissesto idrogeologico. meriterebbe ancora più attenzione di quella che le viene data con l'ultima PAC, al pari di tutte quelle imprese che puntano sulla sostenibilità. cento dei contributi vengono ancora distribuiti in base alla grandezza delle imprese o al numero di animali allevati, con la conseguenza che l'1,8 per cento delle imprese prende il 32 per cento di una torta di 400 miliardi di euro. Nel frattempo anche i teorici della crescita, che dicevano che bisognava puntare sulla produttività e sul mercato globale, stanno ammettendo che la partita è persa. Non riusciremo mai a concorrere con Paesi che hanno *standard* di tutela delle persone, dell'ambiente e degli animali molto più bassi dei nostri. Bisogna allora cambiare strategia, guardando alla qualità e alla sostenibilità, perché questo è l'unico modo che il sistema ha per non fallire. Già da tempo tra i consumatori europei sta maturando una maggiore attenzione. Come dimostrano petizioni e sondaggi, sempre più persone non sono più disposte a tollerare la sofferenza degli animali negli allevamenti intensivi e sono anche disposte a pagare un prezzo maggiore per cibi di qualità. La strategia Farm to fork, con il suo impegno per le piccole imprese agricole e i prodotti regionali, il contrasto alle filiere troppo lunghe e la tutela della salute delle persone e degli animali va sicuramente nella direzione giusta. Le resistenze delle grandi *lobby* agroalimentari contro questo cambio di paradigma nella distribuzione degli aiuti vanno superate. Certo, una trasformazione così radicale aumenterà i prezzi di certi alimenti, ma farà risparmiare sui veri costi. Una cotoletta che costa 2 euro, in realtà la si sta pagando 20 tra costi legati alla perdita della biodiversità, all'inquinamento dell'acqua, al riscaldamento globale, alle maggiori spese sanitarie per un'alimentazione sbagliata. Qualcuno potrebbe obiettare e chiedersi come la mettiamo con le eventuali strategie di *dumping*. L'Unione europea rappresenta uno dei più grandi produttori di cibo a livello mondiale e per evitare la concorrenza sleale basterebbe introdurre una clausola specchio per cui è consentita l'importazione solo di quei prodotti che rispondono agli stessi criteri di sostenibilità. Anche la costruzione di un sistema di facile comprensione circa gli effetti sulla salute dei prodotti alimentari non va demonizzata. Il problema del nutri-score è che misurando solo grassi, zuccheri e sali senza tenere conto degli additivi e dei residui di pesticidi, di pesticidi, non tiene conto del processo di lavorazione quando tutti gli studi dicono che i prodotti ultra trasformati sono quelli più nocivi. Finisce così per costruire una comunicazione distorsiva che non mette al riparo dai prodotti ultra trasformati e non spinge i cittadini ad una dieta equilibrata. Il problema non è infatti il vino o il formaggio, ma quanto se ne beve o quanto se ne mangia. È giusto allora che l'Italia esprima i dubbi rappresentati nella mozione che stiamo per votare, ma ciò deve servire per rafforzare e non indebolire l'impegno per una transizione ecologica che, non dimentichiamocelo, è l'ultimo treno per la salvezza del pianeta. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie.

è da tempo che la strategia Farm to fork sta occupando una posizione di primo piano soprattutto nell'agenda europea. È un progetto indubbiamente importante e di rilievo che però, come è stato ben detto anche prima, rischia di essere compromesso da modelli di etichettatura quali quello del nutri-score che di fatto penalizzano molti prodotti alimentari, tra cui certamente quelli *made in Italy*. A tale proposito occorre quindi operare una premessa; siamo tutti consapevoli del ruolo centrale della nutrizione per il benessere della società, ma non solo, il suo ventaglio di azione è ben più ampio se si pensa al fatto che le modalità di produzione sono centrali nel raggiungimento di un maggiore equilibrio tra l'uomo e le sue attività. Non si tratta affatto di un tema secondario, ma di un tema centrale anche a livello europeo. È proprio in questo contesto che si sviluppa la strategia Farm to fork. Si tratta di una strategia che l'Unione europea insieme a quella sulla biodiversità per il 2030 ha trasformato nel perno del *green deal* europeo, a testimonianza del fatto che ambiente e nutrizione sono strettamente correlati. Una transizione ecosostenibile dei sistemi di produzione, lavorazione e trasporto passa anche e soprattutto attraverso scelte consapevoli dei consumatori. La sfida verde che l'Unione europea si è imposta nel suo nuovo corso e che dovrebbe portarci nei prossimi trenta anni ad ottenere in maniera progressiva un impatto zero sulle emissioni delle attività dell'uomo si sviluppa necessariamente attraverso il ruolo strategico dell'agricoltura e delle produzioni alimentari. Con la strategia Farm to fork si vuole perseguire il conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano. In quest'ottica l'importanza di un sistema alimentare solido e resiliente diventa altrettanto importante e in grado di assicurare ai cittadini un approvvigionamento sufficiente di alimenti a prezzi accessibili. Si tratta certamente di obiettivi ambiziosi, che coinvolgono direttamente tutti i soggetti protagonisti della filiera alimentare, chiedendo loro di trasformare il modo di produrre attraverso soluzioni che comportano una progressiva riduzione di pesticidi e fertilizzanti sui sui campi, ma anche la bioeconomia circolare, con l'uso di energie rinnovabili, produzione di biogas e bioraffinerie, per produrre alimenti per il bestiame partendo dagli scarti di altre lavorazioni. Se si guarda al contesto in maniera più ampia, ci si potrà facilmente accorgere del fatto che proprio la zootecnia italiana ha intrapreso questa strada da anni, con ottimi risultati. Certo si può fare meglio ed è questo l'obiettivo che si è posta l'Unione europea, attraverso una rimodulazione della politica agricola comunitaria, i cui finanziamenti andranno a sostenere branche importanti dell'intero comparto, quali l'agricoltura biologica o l'agricoltura di precisione. È quanto mai importante, dunque, concentrarsi sul come questi obiettivi dovranno essere raggiunti. È infatti vero che la strategia Farm to fork è accompagnata da un cronoprogramma, molto serrato, che prevede interventi da inserire nella legislazione settoriale. Ma è altrettanto vero che, proprio alla luce di queste scadenze, diventa essenziale valutare l'impatto di una simile metodologia sul contesto nazionale specifico. Da qui nascono alcune criticità. Sono numerosi gli studi che hanno dimostrato che tale strategia determinerebbe una sensibile riduzione della produzione agroalimentare, con il conseguente aumento dei prezzi ed un arretramento dei commerci mondiali. Il dibattito si sta però focalizzando su un aspetto specifico, ossia sul modello di etichettatura, che vede appunto due modelli in contrapposizione: quello nutri-score, promosso dalla Francia, e quello, sottolineato prima anche dal Sottosegretario, sostenuto dall'Italia, cioè il nutrinform battery. Nonostante risulti evidente che il secondo modello, quello da noi sostenuto, sia sia più rispondente agli obiettivi di sistema, Francia, Germania e altri Paesi europei hanno progressivamente fatto proprio, invece, il sistema nutri-score, ingenerando una serie di preoccupazioni, almeno per due ordini di ragioni. Innanzitutto, vi è un profilo più strettamente tecnico-scientifico, che riguarda l'effettiva idoneità di questa metodologia, pronta a fornire informazioni nutrizionali e qualitative sugli alimenti, realmente in grado di supportare la finalità di tutela della salute dei consumatori. Ad oggi sembra che questo sistema di etichettatura si basi, però, su valutazioni parziali e fuorvianti, che non tengono in debito conto il giudizio nutrizionale del singolo ingrediente, nel quadro di una dieta complessiva varia e bilanciata, danneggiando così, in primo luogo, proprio lo stesso consumatore. Vi è poi un profilo economico che desta molta perplessità e preoccupazioni. Faccio riferimento al prevedibile impatto negativo che un simile sistema di etichettatura potrebbe generare sull'economia nazionale di Paesi come il nostro, per i quali il comparto alimentare, con le sue eccellenze universalmente riconosciute, rappresenta, non solo una certezza, ma una rilevante componente del PIL. Pensiamo, a titolo esemplificativo, alla proposta dei fautori del sistema nutri-score di inserire una lettera F su tutte le bevande che contengono alcool, anche se in minima parte. Molte economie, tra cui la nostra, ne risulterebbero ovviamente fortemente penalizzate e svantaggiate. Un simile sistema, pur partendo dalla finalità propugnata di perseguire obiettivi di tutela della salute dei consumatori, senza dubbio si traduce in una forte penalizzazione per tutti quei Paesi che, come l'Italia, in ragione dell'elevata qualità e dei livelli di eccellenza della propria produzione alimentare, risulterebbero fortemente competitivi. Il rischio concreto di questo sistema è che la politica economica e commerciale finisca con l'alterare la concorrenza sul mercato, penalizzando alcune economie.

e che - vale la pena ricordarlo - perseguono obiettivi di rafforzamento della coesione economica e della solidarietà tra gli Stati membri. Ecco perché, con questa mozione unitaria, chiediamo al Governo di di intervenire in fretta e bene. È indispensabile che si faccia portavoce dell'esigenza di ottenere valutazioni di impatto approfondite prima che si passi all'attuazione degli interventi del programma di azione. È necessario informare in modo corretto i consumatori, educandoli ad un regime alimentare salutare, in un più ampio quadro di stile di vita sano. In questo le eccellenze enogastronomiche italiane fanno scuola, perché sono la chiara rappresentazione di uno stile di vita sano ed equilibrato. È dunque necessario che il Governo agisca bene e in fretta.

quanto condivisibili vengano annullati da un approccio che, invece di agevolare, finirebbe per penalizzare il mondo agricolo. Questo è il nostro obiettivo ed esprimo

Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, permettetemi prima tutto di ringraziare i colleghi della Commissione agricoltura per il lavoro che abbiamo fatto, e in particolare il presidente Vallardi, per la sensibilità dimostrata nel voler coinvolgere anche l'opposizione nella stesura di un documento condiviso a cui abbiamo aderito convintamente. Non poteva che essere altrimenti perché, quando si parla di interesse nazionale e di difesa dell'interesse nazionale, non abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno e il nostro contributo. La difesa del nostro agroalimentare corrisponde infatti anche alla difesa dell'interesse nazionale, non solo sotto il punto di vista economico, per il grande valore che rappresenta il settore per il PIL nazionale, ma anche perché il nostro agroalimentare è frutto non solo della capacità imprenditoriale di tanti agricoltori, allevatori e trasformatori, ma anche della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Voglio ringraziare anche il sottosegretario Centinaio e il ministro Patuanelli, che non è presente, per l'impegno che stanno dimostrando e per gli sforzi che stanno facendo sia a livello nazionale che europeo per la difesa del nostro *made in Italy*. Mi permetta, signor Sottosegretario, di stigmatizzare anche il fatto che non ravviso e non ravvisiamo lo stesso impegno da parte del resto del Governo o da una parte di esso. signor Sottosegretario, la difesa dell'agroalimentare passa anche attraverso politiche economiche di supporto e valorizzazione del comparto. Non si può - purtroppo, dico - sbandierare il fatto che nell'ultima legge di bilancio le risorse per l'agricoltura sono raddoppiate rispetto alla precedente legge quando in termini assoluti, su una manovra di oltre 30 miliardi, non si arriva che a poche centinaia di milioni come risorse dirette per il settore (naturalmente parlo di risorse dirette). Non si può dire che si crede nel settore se nel PNRR si investono in agricoltura poco più di 6-7 miliardi su un Piano di circa 300 miliardi. Non solo c'è poca attenzione sul piano economico, ma penso anche al sistema bancario, dove i nostri agricoltori, pescatori e allevatori trovano enormi ostacoli per l'accesso al credito. In sintesi, Sottosegretario, nonostante il suo impegno e nonostante l'impegno del Ministro, non ci sembra che il Governo nella sua totalità investa in maniera sostanziale su questo settore, che rappresenta quasi un quarto del PIL nazionale. Così, signor Sottosegretario, non vedo neanche una politica estera che si muove a tutela degli interessi nazionali e a protezione del settore. Penso ad esempio alla pesca (faccio un esempio su tutti), dove non c'è una politica forte a tutela dei nostri pescatori e a difesa dei nostri mari (penso ai rapporti con i Paesi del Nord Africa e con i Paesi dell'Adriatico). Anzi, spesso rappresentiamo purtroppo in questo settore il ventre molle di un'Europa che ha lasciato al suo destino il settore della pesca nel Mediterraneo, difendendo invece a spada tratta la pesca oceanica. E potrei andare oltre. Veniamo invece al tema della mozione. Vorrei sottolineare come sia stato messo in evidenza il modo in cui dobbiamo affrontare la strategia Farm to fork, cioè con pragmatismo, senza lasciarci andare ad entusiasmi ambientalisti spesso ideologici. Lo dico in particolare a quei colleghi che affrontano la questione ambientale senza avere però una visione pratica del problema. Lo abbiamo scritto con chiarezza, riportando studi importanti, come quello del Dipartimento dell'agricoltura americano o del Centro comune di ricerca, che avvertono del pericolo che una strategia spinta del Farm to fork possa creare paradossalmente effetti negativi per la nostra economia. I dati sono chiari: riduzione sensibile delle produzioni agricole europee dal 7 al 12 per cento, a seconda della vastità dell'applicazione di queste strategie; aumento dei prezzi al consumo di circa il 17 per cento; una sostanziale diminuzione delle produzioni e un grosso aumento dei costi, che metterà in difficoltà le nostre aziende; un aumento delle importazioni da Paesi extra-UE, dove i controlli sono assai ridotti, come sappiamo, creando poi quelle condizioni nel resto del mondo (come deforestazione e aumento delle produzioni massive con uso della chimica ancora maggiore) che invece stiamo tentando di arginare qui in Europa. Anche alcune imposizioni, come la destinazione del 10 per cento dei terreni agricoli alla biodiversità, vanno ridiscusse e analizzate in base a principi di costi e benefici. Questa disposizione a mio avviso danneggia ancora di più la nostra agricoltura nazionale, che, a parte situazioni geografiche specifiche, non ha a disposizione vaste quantità di terreno. La morfologia della maggior parte del territorio nazionale ha già di per sé corridoi verdi e aree per la biodiversità e non possiamo quindi applicare questa disposizione in maniera lineare. Penso alle tante zone collinari, dove vi sono numerose coltivazioni, dove il terreno viene usato fino all'ultimo metro e dove peraltro ci sono già zone naturali non coltivate che possono permettere il passaggio o la salvaguardia della biodiversità. Penso all'imposizione dell'aumento del 25 per cento del terreno agricolo destinato all'agricoltura biologica. Ottimo proposito; ma abbiamo il dovere di salvaguardare la qualità del cibo, così come di garantire a tutti la possibilità di alimentarsi con prodotti sani e garantiti. Sappiamo che le produzioni biologiche diminuiscono sostanzialmente la resa del terreno; conseguentemente, ci sarà un aumento dei costi. Personalmente credo che non possiamo creare un'agricoltura tale da dover dividere poi tra consumatori di serie A e di serie B, cioè fra consumatori che possono permettersi prodotti costosi rispetto a consumatori costretti a cibarsi di cibo di scarsa qualità proveniente da altri Paesi. Anche su questo dovremo riflettere e non accettare imposizioni che non tengano conto delle specificità italiane, dove, biologico o meno, vi è un'alta qualità dei nostri prodotti agricoli.

del loro vero apporto in un sistema alimentare complessivo. Tanto è già stato detto su questo e molti colleghi hanno ben spiegato cosa significhi, ragion per cui non mi ripeterò. Voglio, però, evidenziare come per noi sia importante la valorizzazione del sistema nutrinform battery che, in contrapposizione al nutri-score, può dare effettivamente informazioni serie al consumatore per valutare l'acquisto di un determinato prodotto in base alle proprie esigenze alimentari.

e a introdurre anche nuovi sistemi di sperimentazione, anche attraverso la creazione di *app* specifiche per avere più dati ed essere più convincenti verso la comunità europea. Sottolineo anche l'importanza del punto 5, che pochi hanno evidenziato, dove si sollecita l'Unione ad adottare specifiche clausole per impedire l'importazione di prodotti che non rispecchino i criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale: un altare, purtroppo, su cui paradossalmente stiamo sacrificando tante nostre aziende. Da tempo parliamo di dazi di civiltà, ma inascoltati. Molto altro potremmo dire, signor Sottosegretario, ma vorrei invitarla - se mi dà un attimo di attenzione - a porre la massima attenzione nel chiedere il massimo appoggio da parte di tutto il Governo sul rischio che stiamo correndo, insito in questo sistema dell'emergenza formale, che in sede europea si applichino politiche economiche e commerciali oltre che sleali, anche ostili e aggressive, soprattutto nei nostri confronti, che vanno ad alterare la concorrenza del mercato favorendo alcune economie e penalizzandone altre, in netta contraddizione con le finalità fondanti della stessa Unione. Su questo punto, a difesa degli interessi nazionali, della nostra agricoltura e del nostro agroalimentare, ci troverete sempre pronti. Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, quello che il Senato ha deciso oggi di mettere al centro delle proprie attività è un tema cruciale; sicuramente lo è per l'agricoltura e per il comparto agroalimentare del nostro Paese; ma oserei dire che forse lo è ancora di più per la tutela di un modello alimentare salutare e per la tutela di uno degli elementi di stile e di qualità di vita tra i più apprezzati nel concetto stesso di *made in Italy*. Come hanno già detto parecchi colleghi prima, l'Unione europea, interpretando la sensibilità, la disponibilità di dati e di sperimentazioni accumulate in questi anni, e una consapevolezza cresciuta nei cittadini sui temi del cambiamento climatico, della sostenibilità ambientale, del benessere animale, della qualità e dell'impatto dell'alimentazione sulla salute animale e umana, e in generale sull'interazione tra il contesto ambientale e la qualità di vita (quindi, anche di salute) delle persone, ha messo in campo in questi ultimi anni, tra le altre, la strategia Farm to fork e quella per la biodiversità al 2030, e sta implementando il quadro normativo sull'etichettatura dei prodotti alimentari per orientare in senso più ambientalmente sostenibile una transizione dei sistemi di produzione, di lavorazione e di trasporto, accompagnata da scelte consapevoli da parte dei cittadini consumatori. La strategia di cui parliamo persegue obiettivi ambiziosi, come è stato detto prima: una protezione di almeno il 30 per cento delle aree rurali e marine europee; trasformazione del 10 per cento delle superfici agricole in aree ad alta biodiversità, l'incremento del 25 per cento delle superfici coltivate a biologico, la riduzione del 50 per cento dell'uso dei fitofarmaci e del 20 per cento dei fertilizzanti; la riduzione del 50 per cento delle vendite totali di antimicrobici. Tutto questo da raggiungere entro il 2030. Parliamo di prodotti per l'alimentazione che dovranno essere realizzati nel rispetto dell'ambiente, di un ambiente più pulito e più sano, di un utilizzo alimentare più consono e più salutare, per una vita più sana e in un contesto più sostenibile e di qualità di vita migliore. un percorso fondamentale e necessario, ma che richiede una gestione per rendere trasparente e corretto il rapporto tra gli alimenti prodotti in questo contesto di regole il nostro - e i prodotti importati e realizzati con regole e condizioni diverse, non sempre altrettanto garantiti, sicuri e rispettosi. Lo dobbiamo per il rispetto che abbiamo nei confronti dei nostri agricoltori e dei nostri consumatori: sarebbe infatti paradossale darci regole più restrittive e quindi magari, come è stato detto prima, produrre di meno, per poi dover importare prodotti realizzati con minori garanzie e magari sarebbe utile riflettere anche socialmente a chi sarebbero destinati questi prodotti con minori garanzie. Per questo chiediamo di valutare l'impatto e i necessari approfondimenti a tutela e garanzia degli agricoltori e dei consumatori. Per quel che riguarda il perseguimento di un migliore utilizzo e di una maggiore consapevolezza sugli alimenti e sui consumatori, questa trasparenza era già regolata dal Regolamento n. 1169 del 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti, che all'articolo 35 prevedeva, appunto, la possibilità di forme di espressione e di presentazione del campo visivo principale, in modo da aiutare i consumatori a giudicare a colpo d'occhio le caratteristiche nutrizionali essenziali degli alimenti al momento dell'acquisto. Il percorso avviato permetteva una sperimentazione ed è appunto sulle modalità con cui dare attuazione a tale previsione che si è aperto il confronto di cui stiamo trattando oggi, perché i modelli che si confrontano

per tutte le stagioni e per tutte le latitudini, con pochi prodotti validi ovunque, con poche e semplici indicazioni per alimentarsi, dove i prodotti vengono trattati esclusivamente sulla base delle caratteristiche intrinseche, a prescindere dal loro utilizzo formaggio, semaforo rosso; prosciutto, semaforo rosso; vini alcolici, bollino nero - a prescindere dalla quantità e dal contesto in cui vengono utilizzati e consumati. Noi crediamo invece che

di storia, di cultura, di tradizioni, lo stesso riconoscimento UNESCO alla dieta mediterranea sono lì a renderlo plasticamente evidente. Il Il nostro Paese non è per un'alimentazione standardizzata; il nostro è il Paese nel quale ci sono 841 denominazioni di origine, 16 miliardi soltanto di produzione, di cui 10 di *export* legato a 286 consorzi di tutela che ne salvaguardano e ne seguono la produzione, che coinvolgono 200.000 operatori del settore.

altrettanto importanti del cosa consumiamo, anche se siamo consapevoli di avere molto da dire anche sulla qualità intrinseca dei prodotti.

delle produzioni alimentari sono sotto attacco, in nome di una globalizzazione massificata e standardizzata. Questo però è proprio l'esatto contrario della peculiarità virtuosa del nostro modello alimentare. Martin Luther King ha scritto che è sempre il momento giusto per fare una cosa giusta e noi siamo qui non a difendere il nostro modello alimentare e, come diceva giustamente il Sottosegretario, la nostra agricoltura; siamo qui a difendere un'idea di alimentazione e conseguentemente di agricoltura, che pone al centro la qualità, la tutela della salute, della vita, con una maggiore consapevolezza a difesa della salute e delle persone. Per questo voteremo convintamente a favore della mozione in

con un'economia di mercato moderna, dove le emissioni di gas serra saranno azzerate e la crescita sarà sganciata dall'utilizzo delle risorse naturali. Due sono le strategie che giocheranno un ruolo chiave nella trasformazione dei nostri sistemi alimentari: la strategia sulla biodiversità per il 2030

e per l'acquacoltura sempre entro il 2030 e quello di destinare almeno il 25 per cento della superficie agricola all'agricoltura biologica sempre entro il 2030.

presenta una serie di contraddizioni sotto l'aspetto economico, ambientale e sociale, oltre ad una serie di rischi enormi per gli Stati come l'Italia che annoverano, curano, coltivano, allevano ed esportano prodotti d'eccellenza. Secondo uno studio

cali di produzione dal 5 al 15 per cento, con i risultati peggiori per il comparto zootecnico bovino-pollo-suino, oltre che per le coltivazioni di cereali, semi oleosi e ortofrutta. Sempre nel *report* di cui facevo cenno, a fronte di questa diminuzione di produzione è previsto un aumento netto dei prezzi di produzione dei prodotti agricoli di circa il 10 Inoltre, stando a quanto riportano i cambiamenti nella produzione europea, comporterebbero un calo delle esportazioni, nonché un peggioramento del deficit commerciale dell'Europa. Tuttavia, uno dei punti più critici tra quelli prospettati dalla relazione riguarda l'ipotesi degli effetti di questa strategia sulle emissioni. sottolinea come la strategia Farm to fork potrebbe contribuire a ridurre del 28,4 per cento le emissioni di gas ad effetto serra del settore agricolo entro il 2030, ma il *report* mette anche in luce come oltre la metà dei gas serra che l'Europa risparmierà sarà invece prodotta da aumenti equivalenti di gas serra nei Paesi terzi, dovuti proprio all'aumento di produzione agricola di quei Paesi, volto a sopperire al calo

la strategia Farm to fork arrecherà importanti perdite a tutta l'agricoltura europea. La riduzione del 50 per cento dei pesticidi, del 20 per cento dei fertilizzanti e del 25 per cento dei terreni coltivati a biologico entro il 2030

dati allarmanti che in parte confermano l'unico studio di impatto esistente divulgato da United States department of agriculture (USDA). Secondo l'analisi americana Economic and food security impacts of EU Farm to fork strategy, l'introduzione della nuova strategia provocherebbe un calo del 12

Un'altra proposta controversa è quella di introdurre un'etichettatura nutrizionale obbligatoria fronte-pacco che renderebbe il sistema fuorviante e penalizzante per molti prodotti di eccellenza dell'agroalimentare. Parliamo del cosiddetto nutri-score. Si tratta di un sistema di etichettatura dei cibi in cui a ogni colore corrisponde il livello di sostenibilità ambientale di un determinato alimento. Il tipo di calcolo ipotizzato darebbe colori arancione e rosso, identificandoli come scarsamente sostenibili, a molti prodotti della dieta mediterranea. Questo per l'Italia sarebbe un grandissimo problema. Per assegnare un colore a un determinato alimento si usa infatti un algoritmo che andrebbe a penalizzare molti cibi pieni di grassi, dunque molti di quelli apprezzati dalla nostra dieta mediterranea. Pertanto, escluderebbe dalla dieta alimenti sani come l'olio extravergine di oliva, il grana padano, il parmigiano reggiano

più determinata con riferimento alle procedure che orienteranno la politica agroalimentare europea per i prossimi anni, reclamando nuove e più dettagliate valutazioni di impatto e criteri di calcolo equilibrati in merito alle etichettature e che incentivasse la sperimentazione e l'utilizzo, impegnandosi con forza sui tavoli europei per l'alternativa italiana alla nutri-score, ovvero il nutrinform battery che indica la percentuale di energia (grassi, grassi saturi, zuccheri e sali) indicati in grammi presenti in una singola porzione di alimento e il contenuto energetico espresso sia in joule, che in calorie della singola porzione rispetto alla quantità giornaliera raccomandata. Il sistema mette al centro il consumatore e non il mercato globale, valorizza la capacità critica del cittadino che non deve essere fuorviato da colori o immagini che nulla hanno di scientifico e difende quindi il patrimonio unico della dieta mediterranea. Diversamente, si finirebbe solo con l'aggravare la già precaria situazione delle aziende agricole che devono fronteggiare l'aumento dei costi sia delle materie prime, che dell'energia. Questi sono problemi di grande attualità di questi giorni. A loro carico si prospettano nuovi oneri burocratici e costi gravosi, un pericoloso pregiudizio contro gli alimenti di origine animale. I cambiamenti imposti genereranno un prevedibile aumento delle importazioni di questi prodotti alimentari provenienti dai Paesi terzi che non sono soggetti al rispetto di tutti i requisiti in termini di sostenibilità che vengono invece richiesti alle aziende europee e italiane. Esse corrono il rischio di ritrovarsi nella concreta difficoltà di non riuscire a curare le proprie colture per via di una progressiva riduzione degli strumenti di difesa, senza che ci sia, al contempo, alcuna possibilità di accedere a mezzi sostitutivi meno invasivi e nocivi. Sventiamo quindi questo attacco alla dieta mediterranea invasivi e nocivi. Sventiamo quindi questo attacco alla dieta mediterranea che deprezza il nostro *made in Italy* per favorire un livellamento delle abitudini alimentari dei popoli europei a vantaggio dei soliti colossi della produzione e della grande distribuzione. Abbiamo il dovere civico, l'obbligo morale e la responsabilità politica di sostenere e dar forza in questo momento al Governo in questa battaglia di umanità e giustizia sociale, di equità e condivisione, di rivendicazione delle nostre radici, di valorizzazione delle nostre produzioni, di salvaguardia degli agricoltori e delle comunità locali. Il problema è il punto di compromesso; la politica deve tenere conto di quanto è possibile fare per il bene comune, contemperandolo però con quanto è necessario non fare sempre per il medesimo bene

oggi, così come lo scorso 10 giugno, ci troviamo a discutere del nutri-score all'interno del contesto della strategia Farm to fork. Da quel giorno riscontro maggiore consapevolezza nel problema e impegno per la risoluzione dello stesso da parte dell'Esecutivo e del Ministero. Ringrazio i i sottosegretari Centinaio e Battistoni e la nostra capogruppo Bernini per tenere sempre alti i problemi così sentiti. la stessa volontà tra i colleghi della Commissione agricoltura; ringrazio il presidente Vallardi e tutti i colleghi, così come è stato già detto, con i quali abbiamo deciso di portare in Assemblea questa mozione condivisa per dimostrare il nostro costante sostegno nei confronti dell'eccellenza dei prodotti agroalimentari. Un settore che vale ben oltre 522 miliardi di euro. A questo settore, traino dell'economia, traino del nostro PIL e una delle materie prime fondamentali, si chiede uno sforzo non indifferente al fine di raggiungere con successo i tanti obiettivi prefissati. Uno fra tutti la neutralità climatica entro il 2050. È quindi evidente come sia necessario ora più che mai mettere in atto qualsiasi strumento efficace al fine di supportare il lavoro dei nostri imprenditori agricoli, veri e propri custodi del patrimonio naturale italiano. Bisogna farlo per tutelare le produzioni, la nostra competitività in Europa e nel mondo, in un contesto dove la concorrenza, spesso sleale e spietata, sembrerebbe non aiutare il *made in Italy*. Bisogna farlo anche alla luce delle innumerevoli sfide già affrontate dai nostri imprenditori, i quali anche in un periodo di estrema emergenza come la crisi sanitaria hanno dimostrato alti livelli di resilienza, garantendo il cibo sulle nostre tavole quando ciò non era del tutto scontato. Si sono aggiunti inoltre le epidemie di xylella e peste suina, l'eccessiva presenza di fauna selvatica, eventi climatici straordinari, mancanza di manodopera, poche garanzie del reddito dei nostri imprenditori, aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. All'interno delle politiche dei Paesi dell'Unione europea ci si approccia alle problematiche in modo naturalmente differente, ma la sintesi da trovare per regole comuni deve essere necessariamente condivisa e armonizzata tra tutti. Penso alla necessità di scegliere un sistema di etichettatura nutrizionale unico nell'ambito della strategia europea sugli aspetti sanitari connessi ad esempio ad alimentazione, sovrappeso, obesità e lotta contro il cancro. In Italia, patria della dieta mediterranea, che ricordiamo è patrimonio dell'UNESCO e sistema nutrizionale consigliato ovunque perché sano, si è pensato di presentare quale schema armonizzato europeo il nutrinform battery, che ruota intorno alla scelta consapevole del consumatore. Il sistema antagonista, come abbiamo già ascoltato, proposto dalla Francia, è il tanto discusso nutri-score, il quale con la sua etichettatura a semaforo indirizza, nel vero senso della parola, la scelta del consumatore, di fatto condizionandolo. Come Forza Italia, lo scorso 23 novembre abbiamo presentato il nostro piano anti nutri-score, determinati ad evitare la sua adozione a livello europeo, perché lesiva degli interessi italiani e soprattutto perché pericolosa per il consumatore. ricordo ancora, perché è emblematico: il nostro olio extravergine di oliva, cardine della dieta mediterranea, emblema del nutrirsi in maniera sana, verrebbe etichettato come arancione-rosso, mentre una porzione di patatine, fritte con chissà quale olio, utilizzato chissà quante volte in un qualsiasi *fast food*, secondo il nutri-score avrebbe semaforo verde. Tutto ciò è assurdo, quanto pericoloso, perché tale etichettatura non svolge quello che dovrebbe essere il suo unico compito: informare in modo corretto i consumatori, educandoli ad un regime di alimentazione e ad uno stile di vita sano. È di pochi giorni fa la notizia che lo stesso inventore del nutri-score propone una nuova tinta del semaforo: il nero funereo per qualsiasi prodotto alcolico, scatenando polemiche, non solo in Italia, ma anche in Francia, essendo l'Italia, insieme alla Francia, *leader* nel settore a livello mondiale. tutti i prodotti, solo se consumati in eccesso provocano danni all'organismo. Allora da dove proviene la volontà di etichettare qualsiasi bevanda con un tasso alcolemico superiore al 1,2 per cento come altamente dannosa? Credo sia per la voglia di cavalcare l'onda e di presenziare ai *talk show*. Tutto ciò, però, a danno dei tantissimi produttori italiani e non, ma anche dei consumatori, messi in allarme con un sistema di informazione scorretto e poco apprezzato a livello internazionale. Da differenti studi emerge la volontà del consumatore di ricevere informazioni sulla qualità del cibo che si acquista, sugli effetti sulla salute, quindi sull'apporto in termini di grassi, zuccheri e sali rispetto all'assunzione quotidiana. In particolare il nutrinform battery è il tipo di sistema più apprezzato dai consumatori. Mi auguro che con oggi, in attesa della decisione definitiva da parte della Commissione Commissione e auspicandone saggezza e raziocinio, si possa scrivere la parola fine ad un attacco ingiusto a ciò che rappresenta uno dei nostri fiori all'occhiello, cioè i tesori italiani dell'agroalimentare. Condividendo appieno gli impegni che il Governo assumerà per tramite di questa mozione, come appunto la promozione del nutrinform battery, le iniziative per il riconoscimento del valore delle produzioni *made in Italy*, contrastando il fenomeno dell'*italian sounding*, fino al contrasto delle importazioni di prodotti che non rispettano gli stessi criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale imposta ai produttori europei, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, certa che qualsiasi decisione che verrà assunta dall'Esecutivo

Nel 2020 l'Italia si è confermata al primo posto dell'Unione europea a 27 per valore aggiunto dell'agricoltura, con oltre 31,4 miliardi di euro, davanti alla Francia (30,2 miliardi) e alla Spagna (29 miliardi). Sempre nel 2020 si è registrato in Italia un aumento medio del 9,7 per cento dei consumi di prodotto simbolo della dieta mediterranea, come l'olio extravergine di oliva, la frutta, la verdura, fino alla pasta. A guidare la classifica della spesa è la frutta, con un incremento degli acquisti dell'11 per cento; al secondo posto, l'olio extravergine dove i consumi aumentano del 9,7 per cento; a seguire gli alti profitti fatti registrare dalla pasta fatta con grano 100 per cento *made in Italy*. Ricordiamo che la dieta mediterranea è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell'UNESCO proprio per le sue peculiarità, fondate sul consumo equilibrato di alimenti che appartengono alla cultura e alla tradizione millenaria del nostro Paese, che si caratterizza per il suo variegato patrimonio di biodiversità. allora ingiustificato che si lavori a mettere in piedi sistemi che dovrebbero essere caratterizzati dalla giusta informazione ai consumatori per una corretta alimentazione, ma che in realtà sono più che altro condizionati da logiche di mercato spietate che si fondano esclusivamente su interessi economici. Faccio esplicito riferimento a tutti questi sistemi supplementari di etichettatura, studiati e brevettati da agenzie private e che i burocrati unionisti vorrebbero imporre a tutti i Paesi, senza tener conto del rispetto delle tradizioni e delle culture alimentari che da sempre caratterizzano e rendono unici gli oltre cento popoli europei. Anche per quanto concerne il regime alimentare, questa Europa ragiona in un modo sterile e fondato in modo asettico solo e unicamente su quote e misure. il sistema del nutri-score, seppur arriva al consumatore in modo immediato, fornendo in modo semplice l'informazione richiesta con l'utilizzo di colori e lettere, in realtà fonda il suo giudizio sull'elaborazione di complicatissimi sistemi basati su algoritmi che condizionano il giudizio del consumatore, facendo leva soltanto su alcuni nutrienti come il sale e i grassi, senza fare un ragionamento più articolato, fondato sulle giuste porzioni e dosi da assumere nell'arco di una giornata alimentare. Da qui il paradosso di vedere bocciati prodotti quali il nostro parmigiano reggiano e l'olio extravergine di oliva, mentre al contempo vengono promosse bibite gassate e dolcificate: questa è una vera vergogna. Questo sistema sembra non arenarsi davanti a nulla. Dopo la carne e il formaggio, ora è sotto attacco anche il vino, bevanda che appartiene da millenni alla storia non solo dell'Italia, ma di tutta l'Europa. A guadagnarci saranno di fatto i prodotti ultraprocessati e quelli che possono essere riformulati e costruiti in laboratorio per far sì che i componenti rientrino tutti entro i paletti stabiliti dall'algoritmo. In questo modo sarà facile, ad esempio, ottenere un condimento con un nutri-score verde, mettendoci quel tanto di grasso, magari vegetale, da dare sapore senza alzare troppo lo *score*, così come quel poco di sale che basta a stare dentro il limite che farebbe scattare il punto successivo; un po' di proteine che compensino quel pizzico di grasso in più *et voilà*: il *dressing* è servito. Questa non è la dieta mediterranea. Con un cucchiaio di olio extravergine, che avrà un etichetta di colore giallo, un segnale di allerta del nutri-score, si condisce invece un'insalata in maniera più salutare e gradevole. La grande distribuzione organizzata può amplificare il fenomeno e influenzare le scelte. Il rischio è che si promuovono i prodotti più verdi come più sicuri, per far riempire i carrelli di alimenti che potrebbero avere qualità non sempre ottimale. In definitiva, se il nutri-score è stato concepito come strumento per combattere l'eccedenza ponderale, si ritiene che, al contrario, favorisca un incremento del consumo di alimenti ultraprocessati, che appariranno verdi e salutari ma che non lo sono. Inoltre, non focalizza l'attenzione del consumatore sulla porzione di alimento necessaria e non contribuisce ad una corretta educazione alimentare, poiché penalizza alimenti migliori. È notizia proprio di questi giorni che dalla Francia propongono di aggiungere una sesta lettera, la F, associata al colore nero, per classificare le bevande che contengono alcool anche in minime quantità: è gravissimo, se pensiamo che questo è dovuto al fatto che nel vino è presente una piccolissima quantità di alcol, fra l'altro ridottissima (dal 5 al 15 per cento massimo), che gli darebbe una connotazione di pericolo, tale da denunciarne gli effetti cancerogeni. Questa è una vera e propria strategia del terrore che si fonda sul far crescere le giuste paure dei consumatori senza entrare nel merito delle dovute differenziazioni che devono essere fatte fra l'uso e l'abuso di un alimento. Alla luce di questo insieme di evidenze noi riteniamo di grande importanza che la comunità scientifica nazionale, in particolare gli esperti di nutrizione e coloro che si occupano prioritariamente del tema dell'obesità,

di un alimento. Alla luce di questo insieme di evidenze noi riteniamo di grande importanza che la comunità scientifica nazionale, in particolare gli esperti di nutrizione e coloro che si occupano prioritariamente del tema dell'obesità, intervengano nel dibattito che si sta svolgendo a livello comunitario, sottolineando come, sulla base dell'evidenza disponibile, il sistema dell'etichettatura fronte-pacco proposto dal Governo italiano denominato nutrinform battery vada considerato il più appropriato per aumentare le conoscenze nutrizionali del pubblico e dei consumatori e per fornire ai consumatori stessi le informazioni necessarie per affrontare con maggiore preparazione, e quindi probabilmente con un migliore risultato, il tema della prevenzione del sovrappeso e dell'obesità. Il valore della nostra agricoltura, della filiera agroalimentare e della dieta mediterranea non possono essere svenduti per ragioni che nulla hanno a che vedere con la salute e la sana alimentazione. Cito una frase che sembrava banale, ma che oggi ha un valore a mio avviso inequivocabile. Oscar Wilde scrisse: non riesco a sopportare quelli che non prendono seriamente il cibo. Noi, oltre a prenderlo seriamente a tavola, abbiamo il compito di difendere con le unghie e con i denti il nostro *made in Italy*, perché la filiera agroalimentare italiana e i consumatori ne hanno bisogno ogni giorno. Il Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha portato convintamente in Aula oggi questa mozione, insieme alla Commissione agricoltura. Ringrazio il presidente Vallardi e tutti i componenti della Commissione agricoltura, perché insieme abbiamo costruito una mozione importante e unitaria. Voteremo a favore, per ribadire che non lasceremo nulla di intentato per difendere il nostro patrimonio agroalimentare e le nostre eccellenze del *made in Italy*. *(Applausi).*

l'Italia detiene il primato europeo di prodotti agroalimentari certificati a denominazione di origine e a indicazione geografica: 315 prodotti agroalimentari e 526 vini, 841 eccellenze italiane totalmente diverse tra loro, che rientrano nella cultura della buona alimentazione e confluenti a pieno titolo nella dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'umanità. Una Nazione, la nostra, che per conformazione geografica, clima, territorio e biodiversità rappresenta un *unicum* sul pianeta. Grande ricchezza paesaggistica e naturale fanno da cornice a eccellenti produzioni, non per niente riconosciute e apprezzate nel mondo. Un sistema di certificazioni che ben si integra con la strategia europea Farm to fork, il piano decennale predisposto dalla Commissione europea per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Una strategia che intende porre un freno alle alterazioni delle aree rurali e marine, mantenendo una parte di queste aree ad alta biodiversità e impedendo il più possibile contaminazioni causate dalle attività umane, da questa imperante antropizzazione. Entro il 2030 una serie di interventi normativi in area UE avranno l'obiettivo di raggiungere percentuali di protezione ambientale tali da garantire una produzione sostenibile di beni e di accrescere la biodiversità. Per garantire tutto ciò è necessaria anche la sostenibilità degli interventi da mettere in atto. Questi devono essere preceduti da approfondite valutazioni di impatto per prevenire distorsioni e impraticabilità degli stessi: un'azione che infatti può creare difficoltà alle aziende produttive in questa fase di adeguamento e di cambiamenti anche radicali. È per questo che si chiedono misure volte a sostenere gli sforzi economici e strutturali necessari alla trasformazione in atto. trasformazione che interessa l'intera struttura produttiva in quanto si accompagna ad una quasi generale riduzione delle quantità di prodotto per le superfici coltivate, ad esempio, con metodo biologico, e lo stesso vale per gli allevamenti che, per garantire il benessere animale, necessitano di maggiori spazi o della riduzione del numero dei capi; quindi, adeguamenti strutturali importanti che potrebbero essere penalizzanti in ordine alla competitività sui mercati esteri, data la conseguente crescita dei costi dei costi in proporzione alle riduzioni della produzione. Tale situazione che va attentamente valutata in seno all'Europa per non perdere fette di mercato dentro e fuori l'Europa. Per questo, nella mozione in discussione si chiede in sede unionale una clausola a specchio, che permetta, cioè, le importazioni dall'estero solo per i prodotti che rispettino gli stessi criteri di sostenibilità a cui sottostanno i produttori nella UE, i nostri produttori. Di fronte a questo scenario presente e futuro, fatto di precise indicazioni su diversi aspetti della produzione sana e sostenibile, c'è qualcosa o qualcuno che introduce appigli di varia natura per gettare ombre sulla nostra produzione agroalimentare. Uno di questi è rappresentato dal sistema di etichettatura a semaforo di ideazione francese, cosiddetto nutri-score: una semplificazione grossolana che non fornisce informazioni veritiere sul reale valore nutrizionale del prodotto. E, come se non bastasse, arriva l'ultima trovata, che consiste nell'aggiunta di un colore nero alla variopinta etichettatura del nutri-score. Un bollino nero per indicare la massima dannosità per tutte le bevande che contengono alcol, vini compresi, i nostri vini. Come si può notare, è un attacco a tutto tondo verso le nostre produzioni a vantaggio di nuove soluzioni nutrizionali che nulla hanno a che fare con l'apprezzata dieta mediterranea. A bollini colorati si cerca di delegare tutte le informazioni nutrizionali, quando sarebbero meglio configurabili, per una più consapevole scelta del prodotto, attraverso la proposta italiana dell'etichettatura nutrinform battery, che rende il consumatore maggiormente conscio dell'equilibrio esistente per il consumo dei vari alimenti e del peso che questi possono assumere quotidianamente riguardo al proprio benessere. I nostri consumatori vogliono essere più informati non solo sugli aspetti nutrizionali, ma anche su come il prodotto viene realizzato. Vogliamo una cultura nutrizionale che educhi il consumatore a seguire diete più sane e non direzionarlo seguendo colori con uno sterile colpo d'occhio. È intenzione dell'intero sistema Italia far comprendere all'Europa intera le reali qualità degli alimenti, italiani e non solo, che facciano parte della tradizione mediterranea o meno, e del loro giusto consumo. Il *made in Italy* non può uscire indebolito da imprecise e semplicistiche soluzioni cromatiche che ostacolano ciò che è stato riconosciuto buono e sano da sempre.

sano da sempre. Il nutrinform battery rappresenta quella soluzione più equilibrata che incontra le reali esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla salute e alla ricerca di soluzioni innovative di facile reperimento, quali, ad esempio, le *app*, che possono aiutare nella lettura dettagliata di questo sistema sulle confezioni. Un sistema che consentirà di visualizzare un'etichetta molto completa e basata sulle indicazioni Tutto è nella logica di voler difendere il consumatore, i produttori e tutto il sistema, a partire dall'agricoltura. Si richiede, quindi, il massimo impegno del Governo italiano per sostenere l'agroalimentare e il *made in Italy*, destinando risorse del PNRR al contrasto del fenomeno dell'*italian sounding*, ossia la contraffazione di prodotti che vorrebbero sembrare italiani, ma che tali non sono. Altrettanta determinazione deve essere applicata alla valutazione in termini economici della transizione in atto, quindi alla rivisitazione di tempi e modi per attenuare le penalizzazioni non solo per le nostre aziende, ma anche per la competitività del sistema di produzione europeo rispetto al resto del mondo. Per tutti questi motivi, il voto del MoVimento 5 Stelle su questa mozione sarà convintamente favorevole.

Signor Presidente, il Gruppo MoVimento 5 Stelle si unisce al saluto dell'Assemblea al senatore Romualdo Coviello, scomparso il 21 gennaio scorso. Senatore, nonché accademico, per lunghi anni svolse attività di ricerca nel campo dell'economia agraria presso l'università di Bari e della Basilicata, per poi passare all'attività politica come consigliere regionale prima, presidente del Consiglio regionale e assessore regionale all'agricoltura e programmazione economica della Regione Basilicata. Fu inoltre vice responsabile del Comitato nazionale per lo sviluppo agricolo e professore di economia e politica agraria all'Università di Bari. Eletto senatore ininterrottamente dalla IX alla XIV legislatura, fu anche segretario della Commissione per gli interventi del Mezzogiorno, Vice Presidente della Commissione lavoro e sicurezza sociale, Presidente della Commissione bilancio e programmazione economica del Senato e della Commissione affari europei. Fu anche Vice Presidente del Gruppo italiano Unione interparlamentare dal 2001 al 2006; partecipò a missioni dell'UIP all'estero e ai lavori in Commissioni WTO e ONU. Da marzo 2011 fu membro del Consiglio scientifico dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione. Il suo ricordo, Presidente, ci parla di forte impegno politico per la sua terra, la Basilicata. A lui e alla sua famiglia va il nostro saluto. *(Applausi)*. PRESIDENTE. Senatore Lomuti, ci uniamo al suo ricordo.

infantile, istituita dall'OMS per sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sui tumori infantili e per esprimere sostegno e solidarietà ai bambini e agli adolescenti con il cancro, a quelli guariti, a quelli che purtroppo non ce l'hanno fatta e non ce la faranno nei prossimi anni; alle loro famiglie, così duramente colpite e che vivono sofferenze interiori, disagi e difficoltà economiche e organizzative; ai loro *caregiver*, compartecipi emotivamente, ma pronti a dare ogni aiuto ed assistenza per alleviare le sofferenze fisiche e psicologiche di piccoli, grandi eroi. Il cancro infantile ogni anno viene diagnosticato a circa 400 bambini e adolescenti nel mondo; ogni tre minuti sul nostro pianeta un ragazzo muore ancora di cancro, nonostante i miglioramenti delle diagnosi e dei livelli assistenziali, oggi molto più elevati, e la possibilità di nuovi eccellenti approcci terapeutici. Il tema principale della giornata odierna è ribadire la necessità di garantire un accesso più equo ai trattamenti e alle cure per tutti i bambini e ragazzi colpiti da cancro nel mondo, sia nei Paesi più poveri che in quelli economicamente più avanzati. cure appropriate, somministrate con i tempi giusti e da medici e personale sanitario competenti. Diamo radici alla speranza: per celebrare la vita oltre la malattia, inviamo un messaggio d'amore, un melograno da piantare per sostenere la ricerca sul cancro infantile, e indossiamo un nastrino dorato, simbolo universale della lotta al cancro infantile, affinché esso rappresenti un segno prezioso di vicinanza ai nostri bambini e di attenzione al loro futuro. Riconosciamo loro forza d'animo, il loro coraggio, la loro resilienza. Ogni bambino con il cancro merita le cure migliori. oggi centinaia di migliaia di lavoratori con più di cinquant'anni non sono potuti andare a lavorare e saranno lasciati senza stipendio; si aggiungono alle centinaia di migliaia di lavoratori del comparto sanitario, della scuola e della sicurezza che già da mesi non possono lavorare, perché sospesi dal lavoro, e sono senza stipendio. Inoltre, da oggi anche dei nostri colleghi, sia al Senato che alla Camera, come tanti altri lavoratori, non possono esercitare le loro funzioni. Mi riferisco in particolare, alla Camera, a Pino Cabras, il nostro collega di L'alternativa c'è, e qui al Senato ad altri due colleghi che voi conoscete benissimo: Emanuele Dessì e Mario Giarrusso, che oggi non sono potuti entrare.

e questo Parlamento è sicuramente impoverito, perché, per un provvedimento governativo ancora non convertito, il divieto per alcuni parlamentari a mettere piede qua e a far valere il loro punto di vista impoverisce la democrazia di tutta Italia, priva di rappresentanza una parte del Paese e priva tutti noi di un punto di vista che potrebbe essere utile per prendere le decisioni giuste. Per questo vi invito a riflettere e vi dico che il sottoscritto, insieme a tutti i colleghi della componente di opposizione del Gruppo Misto, farò tutto ciò che è possibile per far venir meno queste norme liberticide che dividono il Paese e lo impoveriscono. Non passerà giorno senza che noi vi ricorderemo tutto questo.

Senza entrare nel merito della misura in sé, so che in Parlamento come nel Paese, come nel Governo, ci sono delle sensibilità differenti e io le rispetto tutte. Ci

possa piacere o meno - certe misure restrittive della libertà personale, che vanno addirittura a toccare un diritto costituzionale come quello al lavoro, possono trovare la loro giustificazione.

mi riferisco - e del tessuto imprenditoriale che rischia di chiudere. Possiamo permetterci di lasciare a casa un milione di lavoratori senza stipendio? una riflessione che facciamo all'Assemblea e al Governo. Stiamo attenti noi che siamo i rappresentanti del popolo, perché, se le regole valgono per i cittadini, valgono anche per i parlamentari. Questo deve essere chiaro.

volto a mettere fine a questa discriminazione. Continueremo nella nostra battaglia, ma mi sembra che ormai i tempi siano scaduti. Oltretutto, gli italiani capiscono l'assurdo: fino a quarantanove anni si può andare a lavorare